In data 13 luglio 2020, il Presidente di sezione delegato dal Presidente della Corte dei conti ha inviato la seguente lettera: «Signor Presidente, a norma dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mi onoro comunicarLe che il Collegio previsto dal primo comma, lettera *c)* dello stesso articolo, il 12 luglio 2020, ha eletto Giudice della Corte costituzionale il presidente Angelo Buscema, in sostituzione del presidente Aldo Carosi, che cesserà dalla carica per decorso novennio dalla nomina il 13 settembre 2020. *F.to* Raffaele Dainelli». A nome di tutto il Senato e dell'Assemblea, auguriamo buon lavoro al neoeletto presidente Angelo Buscema.

altro decreto-legge, altra fiducia: da questo meccanismo non si esce. Questa volta però è stato ancora più brutto delle altre, poiché tanto promesso dal *Premier*, come già è stato detto molte volte ieri, tra pochi giorni sarà pronto e decadrà sabato 18 luglio. E così, i 266 articoli che erano presenti sono diventati un po' di più,

che ha spaziato ovunque. Purtroppo però, per quanto si cerchi di riempirlo con questo o quello, ha dimenticato diverse categorie, che ancora non vedono una minima soluzione e una minima uscita da questo stato di crisi importante. L'esame del provvedimento è stato svolto esclusivamente alla Camera

soltanto 52 emendamenti della Lega sono stati approvati e tutti gli altri bocciati o ritirati, perché non avrebbero avuto futuro. Ciò che ha colpito è stata l'incredibile lentezza: pare che il Governo Conte II non tenga mai conto della variabile tempo,

dove c'è stato il momento della verità. Il collega Manca ha preso la parola per dire: signori, i tempi sono questi; non nascondiamoci dietro un dito, possiamo metterci a discutere e votare gli emendamenti, ma sappiamo tutti benissimo che

Dopo questo momento diffuso di contrizione, abbiamo detto: chiudiamola qua, si va senza relatore e la discussione avverrà solamente in Aula.

è una cosa inaccettabile. *(Applausi)*. Ringrazio il presidente Alberti Casellati per l'efficace sintesi che ha usato per definire gli invisibili. Il Parlamento è diventato invisibile nella Costituzione: è una cosa non sopportabile. Se non a noi, che rappresentiamo un'Istituzione, a chi dovrebbe stare a cuore? Aspettiamo che arrivi qualcun altro a farlo o ci mettiamo noi, con un po' di serietà?

susseguiti uno dopo l'altra, con maggioranze sempre meno coese, ma il disegno di questo Governo è chiaro, soprattutto da parte del MoVimento 5 Stelle. Se non c'è rispetto per le persone e per l'Istituzione, non è un problema che vada tutto a catafascio, che si triti e si disfi tutto. La cosa importante è che ci sia l'uomo solo al comando, un regista che decide di rappresentare un *reality*, ovvero una cosa che sembra vera, ma è una finzione. L'uomo è sempre garbato, elegante, ben pettinato e diretto nelle riprese e negli interventi da sapienti inquadrature: solo lui deve spiccare attraverso i TG e le dirette, che - devo dirlo - sono sempre meno seguite, perché sono piuttosto scontate, ma deve comunque apparire come l'uomo del destino. Dall'altra parte - ne abbiamo avuto dimostrazione soprattutto negli ultimi mesi, ma anche ieri - ci sono i bravi di manzoniana memoria, che randellano con le parole ovviamente la Lega, ma soprattutto Matteo Salvini, in un crescendo così scomposto e brutale che a volte sembra quasi che abbiano la bava alla bocca dal livore.

piuttosto di cosa sarà l'Italia nei prossimi mesi ed anni. Se insultate Salvini così brutalmente, c'è solo un motivo: siete terrorizzati dall'idea di andare alle elezioni, perdere e tornare alle vostre vite. Se pensate che gli italiani siano con voi, che problema c'è ad andare ad elezioni? In conclusione, signor Presidente,

Dobbiamo fare cose che abbiano un senso, perché il Paese possa uscire da questa situazione: facciamo in modo che le imprese ed i lavoratori possano fare e riprendere una

la macchina *(Applausi)*. Semplifichiamo, ma in maniera seria, non barocca, come al solito. C'è una sfida che possiamo accettare, ma cambiamo la testa e la prospettiva.

Dare la propria fiducia vuol dire affidarsi e presupporre di lasciarsi guidare da chi dimostra di essere attento, affidabile, leale e sincero, ma soprattutto presuppone un sentimento di reciprocità. Ecco perché non potremo mai darvi la nostra: non siamo tranquilli e men che meno sicuri; sicuri; non si può dare la fiducia a senso unico né a chi non la merita, predica bene e razzola molto male, avendo disatteso ogni proprio principio, tradendo a più riprese le promesse e le parole date. «Mai con il PD», urlavano dai banchi e in TV i 5 Stelle. «Nessuna ipotesi di Governo con i 5 Stelle», affermava il presidente del PD «È un colpo di Stato mettere la fiducia», si sgolava la collega Taverna quando era all'opposizione. Vi siete dimenticati? Noi no e presumiamo nemmeno i cittadini. Non possiamo dare la fiducia a un Governo che non ha mai dato fiducia a tanta parte di cittadini, imbavagliando e non consentendo ai rappresentanti del popolo, che siamo noi, di dare loro ascolto e voce. Questo Governo, a trazione 5 Stelle e con l'avallo di un partito che si dice democratico, ma che vive di fiducia, scardinando lo Stato di diritto, non potrà mai avere da noi la fiducia che si conquista e si guadagna con la sincerità e la coerenza e non si pretende con arroganza e totale mancanza di rispetto, senza consentire replica né proposta. La fiducia invece è ormai la prassi, in prima o in seconda lettura (*tertium non datur*), anche sul provvedimento più importante che deciderà del futuro del Paese, come questo decreto-legge, decreto-legge, che il rilancio ce l'ha solo nel titolo e arriva in Aula al Senato addirittura senza relatore, raccogliendo lo sconcerto e l'indignazione persino del Presidente della Commissione bilancio, collega di maggioranza, che ha chiesto a viva voce che non si ripeta mai più. Dev'essere davvero sconfortante, frustrante, umiliante e triste, anche per la stessa maggioranza, vedersi passare sotto gli occhi tomi e tomi. quello che ci è arrivato dalla Camera: non vi dico quanti sono i tomi degli emendamenti, pieni di proposte, che neanche si sono potuti aprire, ritrovandosi tutti quanti a votare a scatola chiusa. come «utili idioti» (citando Stalin) né «servi sciocchi»; dirò come persone neanche curiose di vedere cosa contenessero quei chili di carta da mandare al macero, ancora freschi di stampa e neanche sfogliati. Oggi vi ribadiamo quindi tutta la nostra diffidenza sfiducia per chi va avanti con i paraocchi, senza rendersi conto che, umiliando il Parlamento, umilia il popolo italiano. Non possiamo darvi la nostra fiducia, proprio per il rispetto che portiamo al nostro popolo e la responsabilità che sentiamo forte per il mandato che ci è stato conferito. Non possiamo darvi la nostra fiducia per rispetto di tutte le categorie dimenticate e di cui siamo la voce: professionisti abbandonati, che non hanno ricevuto fondi; ricevuto fondi; madri, che hanno dovuto lasciare il lavoro per seguire i propri figli, prese in giro da un inutile *bonus baby-sitter* in periodo di pandemia e contagio, né possono lavorare in *smart working*, perché hanno i bambini da accudire; da accudire; dirigenti scolastici, sui quali avete scaricato tutte le responsabilità di una scuola che è stata l'ultimo dei vostri pensieri. Forse sarebbe stato meglio che non l'aveste pensata proprio, se la vostra pensata è quella di affidare la sicurezza della riapertura al commissario Arcuri, "mister mascherine", che non è mai entrato in una classe, sennò saprebbe che la scuola e il distanziamento sociale sono un ossimoro e basta dividere i banchi per garantire uno spazio adeguato, come si fa quando ci sono i compiti in classe. Per fortuna, almeno alla Camera bassa ci avete concesso qualche spicciolo in più per le scuole paritarie che tanto odiate, visto che la libertà vi indispettisce. per rispetto dei docenti non stabilizzati e degli insegnanti di religione dimenticati; del mondo agricolo, cui non avete concesso neanche i *voucher* per far lavorare gli italiani, per i quali non versate lacrime (per non parlare delle piaghe dimenticate, come la xylella, i cinghiali, la cimice asiatica e i disastri metereologici); dei lavoratori, che tra pochi giorni dovranno pagare le tasse, mentre chi non lavora prende i soldi; per rispetto della libertà d'impresa e dei datori di lavoro, che hanno anticipato la cassa integrazione che a molti non è ancora arrivata e hanno messo in sicurezza le proprie aziende e le sedi delle proprie attività usando, tra l'altro, separatori in *plexiglass*, distributori di disinfettanti in plastica e porzioni monouso di alimenti nelle mense, confezionati con imballaggi in plastica. Si tratta della stessa plastica per la quale avete solo rimandato l'odiosa *plastic tax*, al posto di concentrarvi su incentivi strutturali e fiscalità ambientale mirata, senza rendervi conto che, senza gli operatori ecologici e gli impianti e le aziende di raccolta, avremmo rischiato la tragedia nella tragedia. Non possiamo darvi la fiducia per rispetto del settore dell'*automotive*, del trasporto turistico e scolastico privato, dell'edilizia, del turismo, della moda, dello spettacolo e degli eventi, che sono paralizzati, e con loro loro tutta una filiera di attività collaterali; per rispetto di tutti i commercianti, che hanno dovuto abbassare le serrande e ai quali non avete concesso neanche la cedolare secca sugli affitti commerciali. Per rispetto degli artigiani, che non potranno permettersi il credito d'imposta di un ecobonus per l'efficientamento energetico, che ancora manca di certezze nell'attuazione,

istituzionali: neanche nell'emergenza avete avuto l'umiltà di condividere e trovare il tempo per ascoltare chi vi porta le istanze dei territori. Non possiamo darvi la nostra fiducia, perché non c'è un programma: quel programma nazionale di riforme che l'Europa attende non potrà essere solo un libro dei sogni, ma dovrà essere un concreto piano di investimenti, né potrà essere un piano di mero assistenzialismo, basato sulla spesa corrente, per cui il debito non non potrà mai essere saldato. Uscite dalle piattaforme e dagli schermi, parlate alla gente occhi negli occhi e forse capirete che, dietro la grande dignità del popolo italiano, si nascondono drammi quotidiani terribili. Come ho già detto ieri, e concludo,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 e lotteremo perché possa ripartire, ridando al popolo la libertà che gli avete tolto e quella fiducia che, qua dentro, non vi daremo mai.

Signor Presidente, la settimana scorsa, com'è sicuramente noto, abbiamo approvato, con voto pressoché unanime, un nuovo LEA relativo alla cefalea, qualificandola come malattia sociale. Ebbene, devo fare ammenda, perché mi sono dimenticata - imperdonabilmente - di far rientrare fra le nuove patologie il poliformismo,

non so quanti di voi abbiano dovuto studiare 1.000 pagine in cinque giorni. L'Esecutivo ci sopravvaluta, perché negli ultimi tempi è del tutto inutile

il che consentiva di modificarli, stravolgerli e talvolta cambiarne il senso, fino all'ultima stesura. Nel caso dei decreti-legge vale l'esasperazione del concetto, essendo spesso interessati da modifiche in corsa, in forza di meccanismi di decretazione d'urgenza, sopravvenuta prima della loro conversione, ravvisandovi palesi sintomi di poliformismo. Fra le innumerevoli proposte che abbiamo presentato, statisticamente succede che ve ne siano di buone, ma ufficialmente non ne avete accolta nessuna, salvo appropriarvene sempre e solo in parte e senza ammetterlo, talvolta stravolgendone i contenuti, al punto di sviarne completamente l'impianto complessivo, non solo rendendoli di difficile applicazione,

soprattutto per ciò che riguarda il tema dell'analisi e dei controlli. Insomma, non vi è nulla d'innovativo, quando d'innovazione ci sarebbe tanto bisogno. Di conseguenza, conseguenza, in un momento nel quale vi sono risorse che potrebbero essere spese ben pianificando, ecco che allora ci troviamo nella condizione di registrare che

si sarebbe potuto almeno promuovere in norma la facilitazione per la loro rigenerazione

dicendo che non prendere le risorse del MES sarebbe ed è imperdonabile, ma nel piano nazionale di riforma, laddove quantificate il fabbisogno di interventi in 32 miliardi, parrebbe che abbiate preso per buona una ricognizione del 2018, che li spalmava però a tutto il 2045 e non già da spendere in due anni. Da qui la necessità di fare un piano dettagliato di analisi delle reali necessità e dei risparmi

stiamo parlando di qualcosa per cui dovrà essere certo che vi sarà capacità di restituzione istituzionale,

di legge in conversione le nuove regole per la riqualificazione della spesa, in una logica di investimenti post-Covid-19, che tengano tengano conto delle risorse già disponibili, che ricordo sommano a 25 miliardi di euro, comprensivi delle risorse stanziate e non utilizzate per l'edilizia sanitaria, cui si aggiungono gli oltre 8 miliardi di euro previsti in forza dei reiterati, plurimi provvedimenti emergenziali. forte la preoccupazione che si voglia dare libero sfogo a una pioggia di miliardi, da distribuire senza controlli, come è sin qui avvenuto per le risorse già stanziate, senza prevedere misure dedicate a un piano straordinario di recupero dei milioni

Faccio un paio di esempi e concludo. Tutto ciò sistematizzando l'estensione oraria in regime di lavoro ordinario, valorizzando il *know how* competenziale e professionale dei pensionati e dei pensionandi suscettibili di trattenimento volontario

«Gentile professionista, facciamo riferimento alla sua istanza di prestito emergenziale Covid-19 e alla nostra precedente comunicazione in merito. La informiamo che, al momento, non è ancora possibile erogare il finanziamento a lei concesso, in quanto l'ulteriore stanziamento destinato alla copertura degli interessi da parte di Inarcassa è a tutt'oggi all'esame dei Ministeri vigilanti, che dovranno rilasciare il nulla osta a procedere. Non essendo ancora a conoscenza delle tempistiche ministeriali, sarà nostra premura, previa comunicazione, provvedere all'accredito di quanto spettante non appena ricevute le autorizzazioni necessarie. Banca Popolare di Sondrio. Inarcassa».

della lamentela a tutti i costi, della critica a tutti i costi; però noi qui siamo i rappresentanti dei cittadini e siamo la loro voce in quest'Assemblea. Credo quindi che io, come tutti voi, siamo interessati a queste categorie di professionisti e di lavoratori che, nonostante tutto quello che noi discutiamo in questa sede e che il Governo comunica in televisione, poi si trovano di fronte i problemi. Ho visto che c'è qui il sottosegretario Misiani, approfitto della sua presenza e della sua attenzione per sottoporle questo problema, augurandomi che possa velocemente, il prima possibile, risolvere questa situazione. Il decreto rilancio è un provvedimento di mille pagine, dove ci sono alcune cose che possono essere condivisibili. Avremmo anche potuto votarlo se ci fosse stata davvero una dialettica costruttiva tra maggioranza e opposizione, tra Governo e opposizione. Noi abbiamo dato un contributo,

piccolo artigiano, con un'azienda artigiana idraulica, ha avuto il Covid, lui, la moglie e i due bambini, per fortuna sono guariti, quattro mesi che è fermo e non lavora, non sta facendo un solo preventivo e i clienti che dovevano pagarlo a loro volta non l'hanno pagato. Aveva un fido in banca e avendo quattro operai ha anticipato lui la cassa integrazione, utilizzando il fido della banca e mi chiede che cosa facciamo. Mi dice: voi che siete lì a Roma cosa fate? C'è qualche possibilità almeno di spostare il pagamento delle imposte, visto che sento dire in televisione che forse questa cosa avverrà? Cosa Cosa gli rispondo? Dico che non lo sappiamo, vediamo, speriamo. Noi stiamo chiedendo di poter far slittare il pagamento delle imposte previsto a luglio. Quindi le chiedo anche questo. Se dentro questo decreto ci fosse stato quello che abbiamo richiesto, cioè l'anno bianco fiscale e la possibilità di derogare ai versamenti per le imposte, probabilmente avremmo avuto anche un atteggiamento differente nei confronti del Governo. Esempi come quello di Alessandro ce ne sono tantissimi: il barista che ha dovuto anticipare

onorare il pagamento delle imposte e come mai lo Stato non gli dà un po' di respiro e un po' di ossigeno. Mi sembrerebbe anche giusto e opportuno che ciò accadesse, però mi pare di capire che in questo decreto rilancio non ci sia nulla di tutto questo. Nel decreto rilancio ci si aspettava anche, ad esempio, per la rottamazione-*ter* e il saldo e stralcio che le scadenze delle rate, anziché slittare al 10 dicembre, slittassero alla fine del procedimento di rottamazione per riuscire a dare respiro, in modo tale che si recuperassero le rate che non sono state pagate alla fine. Invece così non è stato. è stato. Sarebbe stato utile che in coda all'ultima rata dovuta si potessero pagare queste rate. Poi c'è il tema della notifica delle cartelle che è sospesa fino al 31 agosto. A settembre i contribuenti vedranno ricevere a casa l'avviso di pagamento, dopo un'estate difficilissima e tutto quello che è successo e che è sotto gli occhi di tutti; il 16 settembre c'è una concentrazione di versamenti IVA ed INPS per artigiani e commercianti, quelli del primo trimestre, ritenute d'acconto per i dipendenti, addizionali regionali e comunali, eccetera. Purtroppo, come vede, la situazione è veramente complicata. Non voglio qui essere, come dicevo, l'interprete della lamentela e basta, ma cerco di essere costruttivo e interprete sì delle necessità dei cittadini che qui in quest'Aula rappresentiamo. Poi ci si aspettava che il decreto rilancio fosse anche un primo passo verso quello che è un annuncio del taglio della burocrazia e della semplificazione, ma di semplificazioni qui non ce n'è. Al credito d'imposta per la sanificazione Al credito d'imposta per la sanificazione sono dedicate 41 pagine; al contributo a fondo perduto 55 pagine; al *bonus* vacanze 46 pagine; al credito d'imposta per locazioni non commerciali 33 pagine;

nel frattempo il Paese reale, il Paese che produce, che lavora, registra un calo di quasi il 40 per cento nelle assunzioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Quindi, i sintomi della malattia sono molto seri e molto gravi. Ritengo che si sia persa una grande occasione con questo decreto-legge rilancio, ovvero l'occasione di poter mettere in atto quelle riforme strutturali

però questi 55 miliardi sono stati stanziati sempre con la solita modalità, ovvero *bonus*, sconti un po' di qua, un po' di là, una serie di rigagnoli che perdono efficacia in un momento in cui c'è una vera, profonda, difficoltà di stagnazione economica. In realtà, si poteva anche osare di più se si avesse avuto fiducia negli italiani, negli imprenditori, nei risparmiatori. *(Applausi).* E come si poteva fare? poteva fare? Si poteva anche mettere a disposizione non 55 ma 150 miliardi, e sa come, sottosegretario Misiani? Rivolgendosi ai risparmiatori italiani, alle famiglie italiane. Abbiamo depositato in questo Senato un disegno di legge per l'istituzione dei conti individuali di risparmio, che sono uno strumento utile alla raccolta di finanza da parte dello Stato verso le famiglie, con un credito di imposta al 23 l'azzeramento della ritenuta che si paga sui titoli. Si sarebbe ottenuto un rendimento molto utile, molto efficace e decisamente appetibile per i risparmiatori che, se con i BTP Italia in quattro giorni hanno dato allo Stato fiducia per 23 miliardi di euro, l'avrebbero data a condizione che noi avessimo avuto fiducia in loro. Avreste potuto fare una bella emissione da 150 miliardi; sappiamo che i risparmiatori italiani hanno 5.000 miliardi di liquidità disponibile; avreste potuto dire

Se avessimo potuto dire agli imprenditori, ai lavoratori, a tutto il ciclo della produzione italiana (e anche straniera) che l'Italia dal 2021 avrebbe

accettato. Con questo decreto-legge rilancio dimostrate di non avere fiducia negli italiani, nei nostri imprenditori, nei piccoli imprenditori come negli artigiani, nei commercianti, nelle partite IVA; quindi, noi non abbiamo fiducia in voi.

Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, con grande sorpresa - forse una sensazione che non avrei dovuto provare - ieri ho scoperto che aver messo la fiducia ha privato l'intero Senato della possibilità di intervenire con il minimo delle possibilità di intervento. Una volta si diceva che un ordine del giorno non si nega a nessuno.

di poter intervenire. È come se si fosse rubato a un povero, che è stato già privato di tutte le prerogative del ruolo, anche l'ultima scintilla di ciò che poteva definire i margini operativi reali della collaborazione.

La prima riguarda il grande tema della scuola. Tutti i giorni sentiamo in televisione e leggiamo sui giornali interventi relativi alla scuola. Non voglio nemmeno parlare di ciò che accade con la scuola paritaria perché mi auguro che ci sia presto una mozione con la quale sia possibile, in ogni caso, far arrivare al Governo le nostre istanze,

cento di studenti che non accederanno a scuola o verranno mandati in un teatro o per cui si aprirà una sorta di circo-tenda fuori dalla scuola.

Noi stiamo segnando un punto di non ritorno nella povertà educativa. Un piccolo esempio basta per capire come mai la scuola dell'obbligo viene esclusa dai *test* Invalsi: chiaramente non ci sono le condizioni oggi per valutare persone che che non hanno ricevuto gli stimoli giusti e opportuni per poter dare una valutazione dell'intero sistema. È come dire: siamo un po' più ignoranti e, quindi, molto più poveri.

Ci sono delle proiezioni accessibili a chiunque. Basta pensare alla famosa piramide rovesciata che descrive l'andamento demografico italiano per immaginare che nel giro di quarant'anni - e sono ottimista

Questo è il rilancio Italia che uno si immagina: come posso rilanciare le politiche per la natalità, come posso rilanciare le politiche per l'istruzione, per l'educazione e per lo sviluppo di capacità e competenze?

sogniamo davvero che questa nostra grande ricchezza, sensibilità e cultura, che ha fatto grande l'Europa, trovi nell'obiettivo salute l'obiettivo forte di convergenza. Non lo troverà sul MES, non lo troverà sul *recovery fund*, ma sulla salute può trovare il suo obiettivo convergenza. Per questo motivo, immaginavamo un'azione coordinata tra tutti per identificare che cos'è oggi la salute pubblica. Questo significa, per noi, un investimento nel ripensamento della formazione dei medici. Lo sappiamo tutti che la facoltà di medicina italiana è fortemente sbilanciata in senso ospedalocentrico, ma molto pochi, pochissimi, sono i crediti dedicati alla salute pubblica. Immaginavamo un ripensamento reale delle figure dei medici di medicina generale e non c'è in questo senso. Terzo e ultimo punto: immaginavamo un concetto di salute che tendesse a valorizzare la cronicità, per lo stesso motivo della piramide rovesciata di cui dicevo, e, quindi, la disabilità. Non c'è niente di tutto questo e noi ce ne addoloriamo. Non riusciamo

Signor Presidente, la discussione in corso è una discussione sulla fiducia. fiducia. Io avrei voluto argomentare, quindi, del perché non ci fidiamo. Adesso non so più che cosa dirvi, perché lo ha spiegato talmente bene il collega Siri che dovrò inventarmi qualche cosa, con grande sforzo. Ci proverò, Rammento rapidamente l'argomento del collega Siri. Noi, ai quali il popolo (o, almeno, una parte di esso, che i sondaggi dicono essere piuttosto consistente) si rivolge, non riusciamo a fidarci di questo Governo, perché questo Governo non si fida del suo popolo e non si fida neanche di noi. Che il Governo non si fidi di noi, che siamo i rappresentanti del popolo, è abbastanza evidente nel *modus operandi*. Qui c'è un discorso di metodo, che è stato sollevato da tanti per cui, quindi, basta un accenno estremamente succinto. Stiamo andando avanti, appunto, a colpi di questioni di fiducia su provvedimenti tecnicamente ingestibili da parte del nostro Parlamento. I Regolamenti parlamentari non consentono di fare una lettura accurata, neanche in una sola Camera, di un di un decreto che, allegramente, veleggia oltre i 250 articoli.

almeno noi della Lega dovremmo qui ricordare l'eccellente lavoro che è stato fatto dal presidente Borghi alla Camera dei deputati. Egli è riuscito, comunque,

dell'onorevole Garavaglia e dell'onorevole Comaroli, la Lega ha cercato di arginare alcuni temi che con l'emergenza non c'entravano tantissimo, comunque la si pensi in merito. Mi riferisco al solito tema della *cannabis.* Come pure ha cercato di occuparsi invece di di cui c'era oggettivamente bisogno, anche se sono viste come un potenziale nemico ideologico dall'attuale maggioranza; e in questo caso mi riferisco al tema delle scuole paritarie.

Ci sono però tante cose da fare, quindi è normale che i provvedimenti siano estremamente complessi. Certo, io ringrazio sempre chi avvicina me, che come è noto sono un professorino anche un po' saccente (questo si sa), alla complessità del reale. Essere qua dentro è una cosa bellissima e ci si avvicina alla complessità del reale in infiniti modi, però fa parte della complessità del reale, per esempio, anche la lettera che ho appena ricevuto: "Caro senatore, salve, sono un operaio artigiano di Torino di quarantasette anni, in cassa integrazione dal 15 marzo. Ad oggi non ho ricevuto ancora nulla da parte dell'ente predisposto al pagamento, come molte altre persone. Siete consapevoli della grave situazione di alcune persone? Trovarsi a quest'età a dover chiedere aiuto a parenti e amici, pur avendo un lavoro, ma non ricevendo nulla da parecchi mesi è umiliante è preoccupante. Le chiedo solo una cortesia: se può fare o dire qualcosa a chi di dovere lo faccia". Qui chi di dovere c'è e l'ho fatto. È chiaro che il plurale di

Però, oltre a questo aneddoto, abbiamo anche dei dati sui gravi ritardi con cui i provvedimenti stanno intervenendo. Forse, allora, anziché immaginarsi dei modi barocchi per provvedere liquidità al sistema delle imprese, c'erano alcune cose che potevano essere fatte e che secondo me - io mi rileggo sempre con attenzione i Resoconti stenografici per vedere se ho detto quello che pensavo che pensavo - derivano da un'iniziale sottovalutazione da parte del Governo di quello che sarebbe successo e che quindi sta succedendo. Scusate, non voglio citare me stesso - cosa inelegante - ma insomma, ricordiamo tutti quando a inizio marzo ebbi l'opportunità (e ne approfittai) di suggerire al Governo che, date le circostanze eccezionali, sarebbe stato opportuno fare un *deficit* estremamente alto, uno scostamento estremamente alto, e intervenire in modo estremamente incisivo, perché questo avrebbe permesso di fare poche cose risolutive. Io questo lo dissi prima che la Commissione europea applicasse la *general escape clause,* perché nella riflessione del nostro partito era assolutamente chiaro che quello sarebbe successo. Adesso non voglio dire che noi siamo quelli bravi, perché chiaramente essere professorino, oltre a essere saccente, aiuta anche un pochino a vedere quello che succederà; infatti, non è mica la prima volta che in Europa le regole vengono cambiate, quindi si è in grado di capire quando si andrà in una certa direzione. Lo si sarebbe potuto capire a inizio marzo, si sarebbe potuto fare un intervento deciso che probabilmente avrebbe risparmiato di disperdere attraverso mille rivoli inefficaci quello scostamento che tanto poi alla fine dovrà essere quello che avevamo chiesto noi, perché con meno di 100 miliardi non è che ce la caviamo

però bisognerà pure che cominciamo a guardarci negli occhi e a dirci cosa vogliamo fare di questo Paese. Facendo subito questo scostamento si sarebbero potute fare alcune manovre incisive sul fronte delle qualità che non si sono volute fare spesso per motivi assolutamente ideologici o, peggio ancora, che si sono fatte dopo perché prima non si potevano fare perché le aveva chieste la Lega, quindi ancora una volta per motivi ideologici. Gli esempi sono tantissimi. Io penso intanto che il ragionamento sull'anno bianco fiscale lo si sarebbe dovuto fare, e lo si sarebbe potuto fare, se si fosse capito che in circostanze come queste si poteva tranquillamente pensare anche a un *deficit* del 10-12 per cento - ripeto, in quelle circostanze - perché, come vi dissi all'epoca e come vi ripeto adesso, nel balletto assolutamente assurdo, ridicolo, controproducente e fallimentare delle regole europee del semestre europeo, se ti aprono la gabbia devi approfittarne, perché l'anno dopo quello che conta è se stai scendendo. Quindi c'è un ovvio incentivo a fare immediatamente un forte scostamento. se tu parti dal 14 per cento - dico una cifra assolutamente a caso - e l'anno dopo sei al 13,5 per cento ed hai dei negoziatori un minimo attrezzati culturalmente - e qui non so se nel degrado generale noi ancora li abbiamo, forse sì

e tanti se la fanno sembrare imprescindibile e salvifica, è semplicemente una ricetta per il disastro, perché è un cumulo di regole procicliche, cioè di regole che quando stai male ti fanno stare peggio. Si sarebbe potuto fare quello

(non nel senso del ministro Costa, ma nel senso che ha un costo). Dopodiché, a giugno ce lo ripropongono nel decreto-legge aprile. Nel frattempo, gli imprenditori hanno vissuto in un clima di incertezza. Il tema della fiducia nei riguardi dei nostri elettori tocca anche un altro punto, che è quello delle riforme. A proposito di questa retorica delle riforme, dell'essere costretti da qualcun altro a fare qualcosa che in teoria noi non vogliamo fare: voi gli italiani li dovete lasciare in pace *(Applausi)*, li dovete far vivere. Non c'è bisogno di riforme adesso, ma c'è bisogno di liquidità. E i provvedimenti per fornirgliela alla fine sono quelli che vi avevamo chiesto noi all'inizio. E anche l'approccio, alla fine, è quello che vi avevamo chiesto noi all'inizio. Allora, per favore, se se vogliamo veramente uscirne, cominciamo a cooperare sul serio. Altrimenti l'opposizione dovrà fare l'opposizione. Vi ricordo sommessamente che i numeri per lo scostamento non li avete, e a un certo punto noi vorremmo anche accettare il costo politico di avere la vostra propaganda a reti unificate che dirà che siamo distruttivi, e ricondurre - e qui concludo - tutto entro l'alveo di una normale dialettica democratica. Un Governo, indipendentemente dalle circostanze, propone delle politiche e poi, se hai i numeri per attuarle, le attua; se non ce li ha, se ne va a casa. Quindi o si comincia da ora su un passo diverso, si accetta il buon senso della Lega, gli si dà dignità nel dibattito e lo si valorizza, oppure si va a casa.

un altro provvedimento e un altro voto di fiducia. Ma facciamo un passo indietro: a metà marzo abbiamo avuto il decreto-legge che si è rivelato purtroppo non una cura, ma un piccolo rimedio, un cerotto. La richiesta del voto di fiducia da parte del Governo sul provvedimento cura Italia ha rotto in quel momento il sentimento di unità nazionale che si stava vivendo nell'emergenza provocata dal Covid, ed ha anche interrotto il dialogo, allora aperto, tra maggioranza e opposizioni. il decreto-legge liquidità, annunciato - ricordiamolo - in conferenza stampa molto prima di esistere, e con un grande, eccessivo spazio dedicato a denigrare le opposizioni in diretta televisiva. Si era annunciata una potenza di fuoco che poi si è rivelata purtroppo un accendino, ma soprattutto ha deluso, perché aveva creato aspettative di una liquidità immediata nei conti correnti e nelle tasche degli italiani. Così non è stato e anche quel provvedimento è passato con un voto di fiducia.

ministri; voti di fiducia; annunci roboanti e avveniristici, nel senso di futuribili; promesse senza riscontro; Stati generali convocati e conclusi senza un programma (che arriverà forse a settembre);

sono la realtà della Nazione e la vita quotidiana delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Il Governo non dimostra comune buon senso e percezione della realtà. Ha un suo *storytelling* che racconta un Paese che non esiste, che è in emergenza non domani, ma ieri; una Nazione in cui la cassa integrazione non arriva, le banche non concedono alle imprese i crediti agevolati e il sistema INPS va in *tilt* esattamente quando serviva; un Paese in cui gli imprenditori sono spinti più a chiudere, che a riaprire; il *bonus* professionisti che non c'è o non è dignitoso e il *bonus* vacanze che non è un credito esigibile, ma un anticipo dell'albergatore e un credito d'imposta. il decreto rilancio nasceva per riscattare l'Italia dalla crisi economica drammatica scatenata dalla pandemia: una crisi di domanda e di offerta della quale, stando alle previsioni di ieri della Commissione europea, l'Italia esce peggio di tutti, con un crollo del PIL previsto pari a meno l'11,2

delle famiglie dispone di risorse finanziarie sufficienti per meno di tre mesi. Tre mesi sono esattamente quel periodo di tempo che che voi avete perso per fare questo decreto rilancio di aprile, che però arriva a luglio. Le famiglie (quelle che hanno retto durante il *lockdown*, hanno erogato servizi ai loro componenti e sono stati piccoli centri di *welfare* sussidiario) sono le più dimenticate, specie se numerose.

di risorse, nell'ambito del *recovery fund*, destinate a sostenere le famiglie e favorire la natalità. L'Istat ci avverte che in Italia siamo già oltre l'inverno demografico, in piena emergenza demografica. destinati all'estinzione se non lanciamo un piano di salvataggio per famiglie e natalità. Insomma, nel decreto rilancio ci sono 55 miliardi di euro impiegati male: quasi un paio di leggi di bilancio, una cifra notevole ottenuta anche grazie al nostro voto sullo scostamento di bilancio. Abbiamo fatto questo nuovo *deficit* per questo tipo di *omnibus*? Inoltre, 266 articoli, migliaia di commi, misure che richiederanno 98 decreti ministeriali attuativi e tanto tempo. È un provvedimento infarcito di cose che non servono al rilancio, è questo il dramma. Mance, marchette e *bonus* a termine, pioggerelle senza, a presidio di questo, una visione politica di progettualità e di sistema ed è stato praticamente impossibile, soprattutto al Senato, presentare emendamenti. Questo decreto doveva far ripartire l'economia dell'Italia e per essere efficace doveva farlo in questi mesi di aprile, di maggio e di giugno, ora. Come chiesto da Fratelli d'Italia, doveva essere snello, immediato, per essere efficace, con zero burocrazia, doveva contenere solo misure di rilancio, secondo tre direttrici precise di strategia: difesa dei posti di lavoro, sostegno a imprese e lavoratori autonomi, sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà. E invece no, no, quanto abbiamo chiesto - che non ho il tempo di ripetere - dallo sblocco degli investimenti alla semplificazione delle procedure nel codice degli appalti, alla

bisogna assumerne il costo e poi si può fruire del credito di imposta, quindi è quasi una presa in giro e di fatto non c'è alcuna agevolazione automatica o iniezione di liquidità: in sostanza nessun rilancio per il

che viene dal latino, significa avere fede, confidare in qualcuno o in qualcosa, significa fidarsi, significa anche affidarsi.

una maggioranza che è in quest'Aula, ma che non rappresenta la maggioranza del Paese, fuori da questo palazzo, fuori dai palazzi di una politica impaludata.

al Governo, da questo lato dell'Emiciclo, ci siano persone incompetenti, inconcludenti, incapaci di ascoltare, incapaci di sintetizzare quello che ascoltano in provvedimenti. Pertanto, vorrei chiedere agli esponenti dell'opposizione, che sono cosi larghi di critiche, se esiste un modello, una ricetta, una proposta che in Europa o nel mondo stia avendo successo rispetto ad una crisi che ha delle dimensioni epocali, mai viste dal Dopoguerra ad oggi. Credo che non ci siano queste risposte e che neppure voi le abbiate. In questo momento la cosa positiva che si dovrebbe fare, anche da parte degli esponenti dell'opposizione, è dare realmente un contributo positivo e di cooperazione fattiva. L'impressione a volte, invece, è che si mettano sul tavolo delle proposte per farsi dire di no e poi poter gridare in questo modo dall'altra parte. Io mi auguro che, con i prossimi provvedimenti, si possa realmente arrivare a un a un dialogo e a un confronto che sia maggiormente produttivo. Perché questo avvenga, però, è anche necessario - ho ascoltato le parole del presidente Casellati, ma credo che sarà importante che su questo punto le Presidenze delle Camere facciano sentire meglio la propria voce - che il rapporto tra il Parlamento e il Governo si costruisca in modo tale che il Parlamento possa pienamente svolgere la propria funzione e quindi le due Camere possano pienamente discutere i provvedimenti del Governo, apportando le modifiche, gli aggiustamenti e gli arricchimenti necessari, quelli

non è più possibile fare. Qui si aprirebbe una discussione che non ha a che fare con la fiducia sul decreto-legge rilancio, ma che prima o poi bisognerà sicuramente aprire, e che riguarda invece la necessità di riforme istituzionali, costituzionali e dei Regolamenti parlamentari. Sarebbe ora che le forze politiche si

Su questo mi auguro possa esserci, da parte di tutti, buon senso, senso di responsabilità, coraggio e capacità di affrontare nodi che ormai è necessario affrontare. Per quanto invece attiene alle misure più importanti, che spingono anche il Gruppo Italia Viva a rinnovare la fiducia a questo Governo su questo provvedimento e sull'azione dell'Esecutivo vorrei citare alcuni passaggi che reputiamo importanti e sui quali il nostro Gruppo alla Camera dei deputati, ove è stato possibile intervenire con gli emendamenti, ha dato il proprio contributo.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 qui ci sono numeri e risorse; da qualche parte 55 miliardi saranno pur stati messi, no? Ci sono poi le disposizioni tese a consentire all'INAIL di destinare 200 milioni derivanti dalla vendita di immobili a un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese.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 c'è la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia, così almeno nella prossima legge di bilancio non staremo più a discutere e a litigare per trovare risorse al fine di sterilizzare queste misure tanto problematiche. l'aiuto alle imprese, c'è il taglio dell'IRAP; sapete quanto Italia Viva abbia caro il tema della fiscalità e della riduzione delle tasse e anche con questo provvedimento si è riusciti a ottenere un risultato. C'è il sostegno alle *start up* innovative: se pensiamo al futuro non possiamo non dare sostegno e supporto a chi opera sull'innovazione e con questo provvedimento si riesce a supportare e ad aiutare meglio chi investe in innovazione. Troviamo la promozione delle società *benefit*; c'è bisogno, con i prossimi provvedimenti, di dare un miglior supporto al terzo settore, che ha lamentato alcune richieste non sono state assolutamente ascoltate. Mi rivolgo quindi al sottosegretario Misiani: bene l'intervento sulle società *benefit*, che è stato accolto, ma il terzo settore chiede altri provvedimenti e di vedere le richieste che sono state fatte. Troviamo risorse importanti per un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nelle sue diverse articolazioni territoriali ed ospedaliere, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene all'assunzione di personale. Il ministro Speranza, qualche giorno fa, ci ricordava che in questi mesi sono state assegnate al settore della sanità risorse maggiori di quanto non sia avvenuto negli ultimi cinque anni. È vero, lo esige

consistente. Viene dato, poi, un primo significativo supporto ai Comuni che tiene conto delle minori entrate registrate. Su questo, Sottosegretario, è importante che nei prossimi provvedimenti si faccia la parte che manca. I sindaci e le amministrazioni lamentano di non riuscire

questo primo importante investimento di 3,6 miliardi a favore dei Comuni, però ascoltiamo ancora la voce che si alza da chi è in prima linea come i sindaci e gli amministratori locali e con i prossimi provvedimenti diamo riscontri positivi alle loro richieste. un sostegno, molto più corposo, alle scuole paritarie. È stato annunciato un altro significativo intervento sulla scuola pubblica statale e paritaria e questo è sicuramente auspicabile. poi, di fare un brevissimo passaggio sulla mobilità ciclabile. Spesso sento dire dall'opposizione parole ridicole sulle questioni legate ai monopattini e alla mobilità sostenibile. Lo ribadisco ancora una volta: i soldi appostati con il decreto rilancio sul *bonus* per monopattini, bici a pedalata assistita e altri mezzi per la micromobilità elettrica non sono stati sottratti alle casse integrazioni né ad altre contribuzioni. Sono stati usati soldi delle aste verdi, soldi che non potevano che essere utilizzati per iniziative come queste oppure, in alternativa, sul trasporto pubblico locale. Ora, poiché sapete anche voi che il trasporto pubblico locale,

per il trasporto pubblico locale? No, si è deciso di usarli per la mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile la si sostiene con azioni concrete, non a parole. Ieri sono usciti i dati di FIAB, la Federazione italiana per l'ambiente e la bicicletta:

sui mezzi di mobilità sostenibile è ancora troppo scarso per fare dell'Italia un Paese che ha davvero attenzione alla mobilità sostenibile. Ci sono altri provvedimenti che abbiamo sostenuto ma sul tema abbiamo sostenuto ma sul tema della mobilità sostenibile dobbiamo ascoltare, ancora una volta, i sindaci che ci chiedono di modificare alcune norme del codice della strada. Non è stato possibile farlo con il decreto rilancio. Sarà necessario farlo con uno dei prossimi provvedimenti, anche in maniera urgente. In conclusione, Presidente,

le misure che il Governo ha deciso e che il Parlamento ha migliorato vengono messe a disposizione di famiglie, imprese e cittadini. Potenziamo quanto di buono è stato messo in questo provvedimento e aiuteremo il nostro Paese a uscire dalla crisi.

ricordo che dietro a ogni ritardo di cui si è parlato prima, bisognerebbe anche verificare il motivo per cui non è arrivata la cassa integrazione o il *bonus.*

i fondi erano arrivati, ma non erano stati distribuiti, le aziende non avevano percorso il giusto *iter*. Si preferisce quindi dare la colpa sempre ai soliti noti, al Governo, all'INPS, senza mai andare a vedere nello specifico e, casualmente, ho trovato davvero tanti errori: fondi stanziati, trasferiti. Vedo il Sottosegretario e ho chiesto anche a lui circa i fondi bilaterali dell'artigianato. Sono già stati sdoganati circa due settimane fa, però quei dipendenti ancora non li hanno. È lì che dobbiamo andare a vedere dove sono i problemi. È lì che dobbiamo tutti insieme controllare che effettivamente l'*iter* giusto sia stato percorso. Certo, si fa prima a dire che è colpa del Governo che non fa nulla.

Dico questo perché è davvero facile fare delle critiche. Io credo che l'opportunità che abbiamo in questo momento, sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, sia dare fiducia ai nostri cittadini. Certo che se continuiamo a lamentarci sempre e a dire che non va bene niente, è ovvio l'effetto su chi non conosce i meandri dell'amministrazione. Anche

Signor Presidente, colleghi, Governo, sarei contenta se l'opposizione si limitasse a fare delle polemiche sterili, perché vorrebbe dire che c'è poco da dire.

È un modo veloce con cui il Governo porta a casa i provvedimenti? Secondo me è un modo con cui vuole, forse, evitare delle trappole; ma in questo danneggia, a mio avviso, anche il Paese, dal momento che su questi argomenti il dibattito è necessario.

Vediamo benissimo che le Regioni del Nord-Est, in parte anche la mia, l'Umbria, sono fra quelle che hanno presentato le maggiori richieste di sostegno a fondo perduto. Significa che il motore dell'Italia, che

Abbiamo visto che i settori più colpiti sono - come ha detto anche il Fondo monetario internazionale questa mattina - le piccole e medie imprese e i servizi: commercio, alloggio, manifatturiero, costruzioni, professionisti, viaggi.

quella che per noi è la piccola e media impresa. Noi abbiamo proposto l'idea di un fondo sovrano, su cui è stato approvato un emendamento, ossia un modo di utilizzare i risparmi degli italiani per sostenere le piccole e medie imprese. Ma su questo, a mio avviso, se il Governo avesse fatto un'attenta riflessione, collegandola ad esempio alla revisione del codice della crisi d'impresa, che è importantissimo in questa fase per il piccolo e il medio imprenditore, non avrebbe fatto un soldo di danno

ci sono provvedimenti che colpiscono in modo abnorme, incomprensibile e ingiusto la proprietà immobiliare. Il nostro Paese è fatto di tanti piccoli proprietari che vanno avanti grazie ai loro affitti. Noi abbiamo gli sfratti bloccati, anche se non erano dovuti all'emergenza Covid,

avevano avviato una procedura di sfratto prima del *lockdown* e che adesso si trovano con l'inquilino dentro che non paga (e va bene), ma senza possibilità di cacciarlo e di rimettere a reddito quell'immobile. Il proprietario che cosa fa? Chiede il reddito di emergenza o di cittadinanza? Questo è un provvedimento irrazionale, che non tiene conto che questa crisi pandemica,

che sono collegate anche a quanto vediamo nel nostro Paese, in particolare - come dicevo - nel Nord-Est. Ma è ovvio che noi, in questa sede, non abbiamo avuto il tempo di approfondirlo. La collega diceva che probabilmente noi dell'opposizione non abbiamo letto il decreto rilancio. Guardi che è vero, ma sono talmente tanti gli interventi che parlarne in un dibattito - come abbiamo fatto - praticamente nullo (è la seconda volta che intervengo e non riesco a coprire tutti i temi)

Non è possibile mettere la fiducia su provvedimenti di questa natura, perché rischiamo rifare un brutto copia-incolla delle politiche europee,

cui i rappresentanti del Paese hanno bisogno e necessità di ragionare, perché tutti noi riceviamo sollecitazioni, tutti noi cerchiamo di capire in che epoca siamo e tutti noi cerchiamo di darci una prospettiva. Che ci sia concessa, allora, almeno la possibilità

Signor Presidente, ho sentito da parte di molti colleghi della

per il Paese l'opposizione dovrebbe invece collaborare in modo molto più costruttivo. Benissimo, stiamo parlando del decreto rilancio, quindi dei 55 miliardi. Ricordo a tutti - perché resti ben ben chiaro - che il 30 aprile, quando abbiamo votato lo scostamento di bilancio di 55 miliardi con la risoluzione n. 101, la maggioranza era in Aula con 158 presenti, che non bastavano a garantire lo scostamento di bilancio. *(Applausi).* Quindi, senza i voti del Gruppo Misto, che non ha votato la fiducia al Governo, e di tutto il centrodestra,

Leggete, studiate, guardate i documenti e forse è il caso che qualcuno cominci anche a ringraziare per il lavoro che qua stiamo facendo.

Il nostro onorevole Gusmeroli alla Camera vi ha spiegato - cosa che tra l'altro avevamo fatto anche nel 2019 - che si potevano rinviare dal 30 giugno al 30 settembre 10 miliardi di acconti e saldi IRPEF e IRES, che avrebbero dato respiro naturalmente al mondo delle imprese.

per ragioni di finanza perché l'effetto finanziario connesso al costo figurativo dell'indebitamento dello Stato era solo 1,5 milioni di euro. Pensate: 10 miliardi di di acconti che si possono spostare di qualche mese dando respiro alle imprese con un costo dello Stato di 1,5 milioni di euro, e la risposta è stata no.

per l'aiuto dei nostri cittadini, tanto è vero che oggi avete pressioni da parte di tutto il mondo imprenditoriale che vanno in questa direzione. Una misura che si poteva assolutamente mettere in campo. a categorie soprattutto nel mondo del turismo - uno dei settori più colpiti - piuttosto che dell'agricoltura, dopo il fallimento della regolarizzazione che ha visto pochissime persone

I *voucher* li chiedono le categorie perché non riescono a trovare il personale, a proposito di gente che perde il lavoro e che potrebbe trovarlo. È uno strumento di flessibilità in questo momento; non avete voluto farlo perché anche qui c'è l'ideologia che vi contraddistingue: non ragioni di bilancio, manca la volontà *(Applausi).* Questa è la collaborazione che chiediamo come opposizione, che ci dovrebbe essere da parte vostra. Non è finita, perché anche sulle opere pubbliche bloccate abbiamo chiesto lo sblocco, ma non di utilizzare nuovi nuovi stanziamenti. Il servizio studi della Camera ha messo in evidenza che ci sono 200 miliardi stanziati dallo Stato nel bilancio, che non vengono spesi per le opere perché queste sono bloccate per ragioni naturalmente burocratiche, di autorizzazioni o meno; sulla Gronda manca solo un'autorizzazione. Abbiamo chiesto di sbloccarle, e il risultato qual è stato? Emendamento respinto, non va bene. No. I nostri nonni nel Dopoguerra avrebbero fatto di tutto per sbloccare le opere pubbliche; le avrebbero messe in campo per aiutare a crescere il Paese e, invece, qua stiamo ancora con i veti incrociati: quest'opera non si fa; quest'altra neanche; c'è il comitato del no. Anche questo è un errore politico e strategico notevole. È una questione che dobbiamo mettere in evidenza perché nel decreto rilancio non ci sono ma anche interventi positivi - lo riconosciamo - come il taglio dell'IRAP, il contributo a fondo perduto, i soldi per la cassa integrazione, però il ruolo dell'opposizione e della minoranza è mettere in evidenza alcuni errori che la maggioranza ha fatto non accogliendo le proposte che la minoranza ha messo in campo. Questo è il nostro dovere.

in gergo ragionieristico. È semplicemente una volontà che non avete avuto e con il passaggio dei sindacati abbiamo allungato i tempi della cassa integrazione. C'è poi qualcuno che dice che i tempi sono lunghi perché le regole e i tempi della cassa integrazione

relativa, effettuare il *login* e fare la richiesta del *bonus*. Quando verrà comunicato l'esito positivo, la richiesta va confermata; poi bisogna attendere la generazione di un QR che dovrà essere comunicato alla struttura alberghiera al momento del pagamento, sempre che questa lo accetti. L'albergatore, a sua volta, dovrà mettere in campo altre procedure: prima di applicare lo sconto, deve accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate con le proprie credenziali e verificare in tempo reale l'ammontare del *bonus* residuo.

*code* e *login* avete escluso tutta la popolazione anziana, quella naturalmente più fragile e che ha più difficoltà ad accedere alle tecnologie. È davvero un ottimo lavoro. Vogliamo parlare dello *stop* alla limitazione del contante? Anche questo costava?

come la possibilità di pagare in contanti rimanga particolarmente importante per taluni gruppi sociali, ad esempio, gli anziani. Il contante, sempre secondo la BCE, è una forma di pagamento ampiamente accettata e rapida, l'unica che non consente legalmente di imporre tariffe per il suo utilizzo e che non richiede un'infrastruttura tecnica. Anche

si favoriscono le organizzazioni criminali. Lo dice la Procura nazionale antimafia. Saranno loro che presteranno i soldi e faranno da usurai alle imprese perché lo Stato non riesce ad arrivare. bisogna contrastare e combattere le mafie e le organizzazioni criminali. Insomma, tutti questi provvedimenti mettono in campo il fatto che l'opposizione ha messo in evidenza degli aspetti assolutamente importanti, che potevano essere accolti e potevano dare quella scossa importante dal punto di vista economico, visto che l'Istat ci ha detto che un'azienda su tre, per il Covid, rischia di chiudere. E se chiudono le imprese, lo Stato non avrà gettito e, senza gettito, non riuscirete neanche a difendere il vostro reddito di cittadinanza e il vostro reddito di emergenza. Senza le tasse che le imprese pagano, non riuscirete più neanche ad avere i soldi per pagare i dipendenti pubblici. Quindi, in un modo molto più intelligente e furbo, se fossi in voi, aiuterei le imprese. Se l'economia va bene, mettete in sicurezza anche le vostre misure, cui tenete tanto. Siete anche poco furbi da questo punto di vista.

capisco, ma non si può parlare di collaborazione tra maggioranza e opposizione se non si mette da parte il risentimento che il MoVimento 5 Stelle ha nei confronti soprattutto della Lega. Io lo capisco, lo comprendo, la politica è fatta così. Mettetelo da parte, però, e magari si riuscirà a lavorare tutti insieme

- vorrei partire da dove ha terminato il collega Romeo, per rassicurarlo che noi non abbiamo alcun tipo di risentimento nei confronti della Lega. *(Applausi)*. In realtà, il risentimento io lo rilevo nelle sue parole, quando dice che avremmo dovuto nominare dei commissari. I commissari sono stati portati avanti, come proposta normativa, dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega nel decreto sblocca cantieri. La lista delle opere da commissariare era pronta ed è la Lega che non ci ha consentito di portarla avanti. *(Applausi)*: opere importanti per il Paese e, invece, la Lega si è fissata sull'opera principe per litigare col MoVimento 5 Stelle. Poi, dopo il Papeete, abbiamo visto che cosa è successo qui ad agosto Per noi le opere importanti sono quelle utili agli italiani. Bisogna parlare di analisi costi-benefici e non di prese di posizione. L'elenco delle opere da commissariare, come altre importanti per il Paese, infrastrutturali,

ma quello è il passato: noi ci stiamo muovendo verso il futuro. Il decreto rilancio è fondamentale, perché sta rifinanziando e potenziando il decreto cura Italia. Ha trovato coperture per le garanzie pubbliche, per il decreto sta intervenendo a sostegno di impresa, lavoratori, studenti, sanità, Forze dell'ordine. *(Applausi)*. Sono tanti i soldi che stiamo mettendo per il mondo delle imprese. Sappiamo bene che si parte da lì, ma non si può contestare il reddito di emergenza per chi non può mangiare.

e a chi fa lavori strutturali di miglioramento antisismico (quindi riduzione del rischio sismico) un incentivo pari al 110 per cento del costo dei lavori. Questo sembra un aspetto secondario, ma è invece fondamentale, perché incidiamo sulla cedibilità del credito d'imposta e sulla sua immediata messa in circolazione. Questo significa che diamo liquidità sonante alle imprese e tutti ormai lo sanno. Le stesse banche stanno facendo comunicazioni a mezzo stampa con cui si dichiarano disponibili a supportare qualsiasi tipo di costo e, quindi, compreranno quei crediti, tanto dal proprietario dell'abitazione o dai condomini, tanto anche dalle imprese di costruzioni o dai fornitori o dai liberi professionisti. Si tratta

al sottosegretario Fraccaro che lo ha portato avanti. È una misura del MoVimento 5 Stelle ed è fondamentale, perché ci consente di guardare a una delle nostre stelle polari: l'ambiente.

La media è di 3,5 miliardi all'anno negli ultimi venti anni. Di questo stiamo parlando. Sono soldi con cui si va a incidere direttamente, perché il cittadino che vorrà costruire e realizzare interventi di miglioramento sismico potrà farlo a costo zero, perché trova un'impresa o un investitore o una banca

esiste una misura di rilancio più proattiva di questa, grazie alla quale l'impresa a costo zero può anticipare i lavori al proprietario e venderli alla banca? Più aiuto di questo? Parlate delle piccole imprese. Ebbene, nel lavoro, soprattutto quello privato, la piccola impresa può tranquillamente subappaltare da un imprenditore più grande; può trovare il suo finanziatore e il suo intermediario finanziario; può andare dalla sua banca;

E poi vedremo quando partirà e ripeto che è notizia di questi giorni che le banche stanno dando la loro disponibilità a comprare il credito. In ultimo, l'aspetto più importante del superbonus, che per la prima volta torna al centro del dibattito parlamentare, è la giustizia sociale: fino ad oggi chi si è potuto permettere di fare lavori di efficientamento energetico o miglioramento sismico? Chi ha i soldi. Oggi, invece, diamo la possibilità anche a chi non ha i soldi di poter compiere questi lavori, di pagare meno la bolletta e soprattutto di avere una casa più sicura.

il riconoscimento del superbonus ai lavori di demolizione e ricostruzione. Molte volte, per migliorare sismicamente un edificio, non bisogna per forza intervenire sull'edificio costruito, ma è meglio abbatterlo e ricostruirlo. questo lo si farà grazie alle competenze degli ingegneri e degli architetti, dei tecnici italiani, che decideranno cosa sarà meglio fare: se abbattere e ricostruire o se intervenire sul costruito. Badate che abbattere e ricostruire significa normativamente adeguare quel fabbricato alla normativa antisismica: palazzi più sicuri *(Applausi),* una casa che varrà di più per il cittadino che, se ha realizzato lavori di efficientamento energetico, pagherà - ripeto ancora una volta - di meno le bollette e magari le azzererà. Secondo punto importante: il riconoscimento il riconoscimento del credito di imposta e la messa in circolazione immediata a stato avanzamento lavori. Non bisognerà più aspettare che finiscano i lavori, ma l'impresa e i professionisti potranno cedere quel credito immediatamente.

iniziamo a lasciarci un po' alle spalle la straordinarietà e pensiamo finalmente alla ordinarietà. Era ora, perché intervenire in ordine ai terremoti in questo Paese significa iniziare a concepire l'ordinario.

Signor Presidente, il Covid ha mandato in soffitta il Patto di stabilità e dal neoliberalismo si sta tornando alle teorie keynesiane sull'interventismo economico. La salvezza viene vista nella maggiore capacità di spesa per alimentare la domanda di beni e servizi. Siccome in una situazione di crisi i privati tendono a risparmiare e le imprese a non investire, rimane solo lo Stato, che torna così ad avere un ruolo decisivo; e lo è ancora di più se si pensa che il crollo dell'economia si è già tradotto in un peggioramento delle condizioni di vita materiali. Come ricordano Banca d'Italia e Istat, un terzo delle famiglie italiane ha riserve finanziarie per tre mesi; un terzo delle piccole e medie imprese è a rischio fallimento; il 40 per cento delle famiglie che hanno contratto un debito è in grado di onorare le rate del mutuo; nell'alberghiero e nella ristorazione, più di metà delle imprese sta affrontando una situazione di estrema criticità. Questo provvedimento si inserisce nel quadro di misure per tamponare l'emergenza cominciato con il decreto-legge cura Italia e con il decreto-legge liquidità. Pertanto, è naturale che contenga alcune misure assistenziali: se la crisi non viene affrontata come una questione sociale, rischia di allargarsi la forbice delle diseguaglianze e colpirà prima di tutto le famiglie numerose, le donne e i giovani. Allo stesso tempo, il provvedimento contiene misure volte a incentivare i consumi e gli investimenti. È giusto incentivare acquisti che vanno nella direzione della *green economy*, come il super *bonus* per le ristrutturazioni ecologiche e gli impianti fotovoltaici. Si tratta di una di quelle misure *shock* che possono dare impulso all'economia: non solo favorisce l'edilizia, ma aumenta anche il valore delle proprietà immobiliari e aiuta l'emersione del sommerso. Bene anche il *bonus* biciclette e monopattini e quello per la rottamazione delle vecchie automobili per indirizzarsi verso la conversione ecologica, assai importante per il bilancio e la ripartenza europea. Convince l'idea di uno Stato che sollecita consumi ambientali sostenibili e scoraggia quelli che non lo sono. La rimodulazione dell'IVA di cui si è parlato nei giorni scorsi dovrebbe servire anche a questi obiettivi. Anche il *bonus* vacanze è una misura giusta a favore delle famiglie e nel dare sostegno all'intera filiera turistica. Bisogna però fare in modo che lo Stato rimborsi in tempo reale le strutture che accordano lo sconto, per evitare che queste si trovino a fare da cassa con ulteriori difficoltà dal punto di vista della liquidità. Ci saremmo aspettati qualcosa di più a favore dei liberi professionisti, perché la proroga del termine al 20 luglio per gli adempimenti fiscali è davvero poca cosa per chi ha gravi problemi di liquidità.

sono state intraprese, ne vorrei aggiungere un'altra. In Germania e in Austria, nella fase emergenziale, l'opposizione ha sostenuto il Governo, cosicché

Tra gli interventi previsti ve ne sono alcuni con ricadute molto positive sui nostri territori. Di particolare efficacia è - ad esempio - l'estensione della rete di gas naturale nelle zone più svantaggiate dal punto di vista climatico. Il provvedimento prevede inoltre che nei territori di montagna le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi si estendano anche agli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente. In conclusione, mettiamo oggi il tassello che garantisce un'uscita ordinata dalla fase del *lockdown*. Con il decreto semplificazioni e l'accordo europeo deve cominciare il secondo tempo della questione economica e sociale, quella per cui l'Italia mette in campo una forte programmazione, in grado di liberare le energie per una ripartenza che sia non solo numerica, ma anche qualitativa. Non dimentichiamo che per una ripresa economica ci vuole sempre la fiducia degli attori principali (cioè le imprese e i consumatori privati); una fiducia che questo provvedimento prova ad alimentare. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

pronunciando la famosa frase per cui noi siamo ormai diventati gli invisibili della Costituzione. La ringraziamo perché sta difendendo le prerogative di questo Parlamento

a tutti, quindi, come questo Governo e la sua maggioranza abbiano come strategia di fondo quella di operare affinché una delle due Camere possa in qualche modo lavorare sul provvedimento riducendo quindi ad un'appendice, ad una mera formalità il bicameralismo perfetto previsto dalla nostra Costituzione. ad approvare con un voto di fiducia un provvedimento, ma è una fiducia che sta tradendo non solo queste Aule del Parlamento, ma anche

di fare. Avremmo potuto - come si dice in gergo - ribaltare i tavoli delle Commissioni e invece ci siamo seduti pazientemente, perché era nostro dovere tentare di modificare il provvedimento. Ed è per questo che voglio ringraziare i nostri colleghi di Fratelli d'Italia della Camera e il nostro presidente Giorgia Meloni, che hanno guidato in quella sede parlamentare delle battaglie cruciali

La questione non è che a me non piace. In questo momento la Presidenza del Senato la sta invitando a rispettare la dignità di quest'Aula. misure inutili che state per approvare, prendendo a riferimento quello che invece ha fatto Fratelli d'Italia, approvando una serie di emendamenti, nell'altro ramo del Parlamento, tra cui l'aumento del 100 per cento e quindi il raddoppio delle pensioni di invalidità agli invalidi civili. Ci siamo però trovati a discutere anche di altre misure che non abbiamo condiviso, perché non c'entravano nulla in questo decreto, gli incarichi di consulenze professionali al Ministero dello sviluppo economico; gli incarichi professionali al Ministero dell'economia e delle i monopattini; le sanatorie per gli immigrati; le nomine nei consigli di amministrazione e perfino i voli in *business class* all'Expo di Dubai che - anche in questo caso grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia - siamo riusciti ad eliminare. Su questo non siamo scesi ad alcun tipo di compromesso né con il Governo, né con la maggioranza, perché quando ci è stato proposto di poter utilizzare come forze di opposizioni delle risorse importanti, fino a un miliardo di euro, abbiamo rispedito al mittente

Signor Presidente, noi avremmo voluto parlare di altro. Avremmo voluto parlare di imprese, di fisco, di aiuti alle famiglie, di tutela dei posti di lavoro. E voglio parlare di alcune proposte, perché i colleghi di maggioranza ci hanno accusato di fare demagogia. Quindi, voglio fare alcuni esempi di ciò che ha proposto

che, con qualche milione di euro, si sarebbe potuto differire il termine per il pagamento delle tasse da parte delle imprese italiane. Queste sono le proposte che voi avete letteralmente bocciato. Così come avete bocciato le proposte che consentivano alle imprese che non mandavano in cassa integrazione i propri dipendenti di avere un contributo in egual misura rispetto a chi invece li mandava in cassa integrazione, per ridurre il cuneo fiscale e quindi il costo del lavoro, che è la vera emergenza è oggi esistente nel sistema Paese. Avevamo chiesto liquidità per le imprese e per le famiglie italiane. Voi avete approvato un decreto liquidità che abbiamo ribattezzato decreto salva banche, che, invece di sostenere le imprese, ha risolto il problema dei crediti incagliati delle stesse banche. Inoltre, avevamo chiesto di eliminare tutte le misure inutili cui ho fatto riferimento poco fa. Signor Presidente, l'aria che si respira fuori da queste Aule è molto pesante. Nel corso delle audizioni che abbiamo svolto nelle ultime settimane presso la Commissione bilancio è stato detto, in tutti gli interventi delle istituzioni nazionali, che il 60 per cento delle famiglie non arriva a fine mese.

a Villa Pamphili, tenendo il Paese bloccato dieci giorni, senza produrre nulla di concreto e di positivo per il Paese stesso. Infatti sugli Stati generali è caduto completamente il silenzio. silenzio. Sono due mesi che aspettiamo il decreto semplificazioni, che ad oggi ancora non arriva, e sappiamo che il ministro Gualtieri è pronto a portare in queste Aule un ulteriore scostamento di 20 miliardi.

morire e fallire moltissime imprese. Sa perché le dico questo? Tentare questa operazione all'inizio sarebbe stato diverso rispetto a ciò che sta accadendo oggi. Voi avete fatto del mero assistenzialismo, che in parte è servito, perché ha avuto sicuramente natura risarcitoria; ma non c'è stata mai la possibilità di avere una visione d'insieme di quello che è stato il sistema Paese. E ci auguriamo che questa sia l'ultima volta che vi sentiremo chiedere il voto di fiducia. Ci auguriamo che abbiate anche la decenza di riconoscere il fallimento totale di questa esperienza di Governo. Mentre qualche vostro giornale amico vorrebbe che contro Fratelli d'Italia fossero usati i fucili e magari vorrebbe vederci tutti appesi a testa in giù, noi continueremo a chiedere libere e democratiche elezioni, perché secondo noi l'Italia merita ben altro: merita un Governo solido, forte, coraggioso, capace di farla tornare a correre e di restituirle quella grandezza che ha avuto. Noi siamo l'Italia, siamo un Paese che merita di essere guidato da un Governo all'altezza della situazione. Per questo Fratelli d'Italia non darà mai un voto di fiducia a questo Governo. *(Applausi)*.

l'Europa, con le deroghe al Patto di stabilità e crescita e sulle regole relative agli aiuti di Stato, ha reso possibile l'esistenza del decreto cura Italia e del decreto rilancio moltissime risorse. Il decreto rilancio sfrutta, fino all'ultimo euro, tutti gli scostamenti, i margini del saldo da finanziare, del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto che il Governo ha chiesto al Parlamento e che il Parlamento ha autorizzato. L'indebitamento netto sale di ulteriori 55 miliardi, dopo i 20 del decreto cura Italia. Sono 75 miliardi di risorse a sostegno del salvataggio dell'Italia. Sono 75 miliardi di risorse che costituiscono maggior debito. Ormai lo dicono tutti: è un maggiore debito a carico dei nostri figli, a carico del loro futuro.

si dovrebbe anche avere uno sguardo di insieme che tenga conto di tutto. Prima la senatrice Unterberger ha parlato di buone prassi che a livello europeo esistono e sono possibili tra maggioranza e opposizione. Sarebbe quindi auspicabile che, nei prossimi passi, anche il Parlamento italiano copiasse tali buone prassi. 75 miliardi sono stati approvati, per quanto riguarda il decreto cura Italia, prima dal Senato e, per quanto riguarda il decreto rilancio, dalla Camera. L'altro ramo del Parlamento ratifica. È stato più volte stigmatizzato in questa sede, ma il monocameralismo è davvero disfunzionale e non rende neanche giustizia ai veri riformisti istituzionali che invece avrebbero voluto un Parlamento molto efficiente. Allora, da questo punto di vista, Presidente, anche immaginare una modifica dei regolamenti potrebbe essere molto importante da qui in avanti. I 75 miliardi sono stati accordati con il voto delle opposizioni, perché gli scostamenti sono stati votati all'unanimità,

l'impossibilità da parte dei professionisti ordinistici di utilizzare il fondo perduto. Non lo dico relativamente alle risorse, perché sono professionisti abituati a fare del loro talento la risorsa per il futuro proprio proprio e della propria famiglia. Ma penso che oggi l'Italia avrebbe bisogno di prendere ad esempio le persone che si impegnano, che studiano e danno risultati con merito. Sarebbe un esempio molto significativo.

È veramente il momento in cui la pubblica amministrazione può dimostrarsi *partner* delle imprese e delle famiglie. Da questo punto di vista, leggendo il decreto rilancio e vedendo la proroga fino al 31 dicembre del 2020 della poi *smart working* non è, è un *home working* - risulta un modo strano per dimostrare la corresponsabilità tra pubblico e privato e forse, invece, è un modo per marcare ancora di più il solco che esiste tra garantiti e non garantiti.

poste in essere misure fondamentali: dalla riduzione dell'IRAP all'abrogazione del saldo 2019 e del primo acconto 2020, il contributo a fondo perduto, il credito di imposta per i canoni delle locazioni commerciali, per i costi sostenuti per fiere poi non realizzatesi, gli incentivi per le *startup,* il virtuosissimo contributo per i dipendenti delle aziende in crisi che decidono di intraprendere una loro iniziativa portando avanti l'*expertise* di quella azienda. Moltissime risorse sono state anche destinate alla parte fiscale, e cito l'ampiamento della possibilità di compensazione: si è già compensato non in quota indebitamento netto, ma comunque si è già compensato, e sono state citate le sterilizzazioni delle clausole di salvaguardia IVA. risorse molto importanti sul lavoro: oltre 18 miliardi di indennizzi e di cassa integrazione. Forse qui si poteva dare un'apertura. Se vogliamo parlare di lavoro in termini transitivi, dobbiamo parlare di chi lavora e di chi dà lavoro. Allora da questo punto di vista, forse il decreto avrebbe potuto iniziare a parlare di decontribuzioni, di riduzione ulteriore del cuneo fiscale, di rimodulazione delle aliquote, di incentivi per l'assunzione soprattutto per i più giovani e per le donne che si trovano particolarmente in difficoltà. Si farà con il prossimo scostamento e naturalmente con la riforma fiscale. Ulteriori risorse, pari a 2,7 miliardi, sono a favore del turismo. Ne erano stati annunciati 4, ma probabilmente ne serviranno molti di più, perché il turismo è uno dei settori Grazie la riduzione della tassa occupazione del suolo pubblico, così da permettere a tutti i ristoratori di ospitare all'aperto, e il ristoro per i Comuni della tassa di soggiorno non introitata sono misure particolarmente virtuose. virtuose. Sono 266 articoli ricchi di spunti molto interessanti. Qualcuno parla a questo punto di interventi a pioggia. A onor del vero, ancora non si intravede una strategia di politica industriale chiarissima, ma una terra economica arsa dal *lockdown* sanitario aveva bisogno di un moltissimi centimetri di pioggia.

e la disoccupazione al 12 per cento, certamente bisogna immaginare di portare ulteriore acqua a questo territorio economico particolarmente arso.

del provvedimento, pur nella consapevolezza dei suoi limiti di metodo e di merito, essendo però perfettamente consapevole delle enormi difficoltà che stiamo affrontando rispetto a un Paese che già era enormemente in difficoltà; talvolta inefficiente, talvolta troppo burocratico e talvolta anche perso - come abbiamo visto ieri pomeriggio in Assemblea - in battaglie ideologico lessicali veramente irrilevanti per i problemi che dobbiamo affrontare qui e anche per i problemi che hanno i cittadini fuori. fuori. Italia Viva voterà sì al decreto rilancio e voterà sì ai prossimi passi importantissimi, piano nazionale delle riforme, *in primis,* perché esso è contemporaneamente una sfida che l'Italia non può più permettersi di non vincere e anche la condizione indispensabile per accedere a quei fondi del *next generation* EU di cui tanto si parla. se non facciamo il piano delle riforme, non arrivano le risorse europee perché l'Europa è cattiva. No, semplicemente questi si chiamano fondi per le prossime generazioni; non si chiamano fondi da spandere e spendere in rivoli senza un progetto per il futuro. Quindi per noi stessi, per il nostro bene e per il futuro dei nostri figli, di cui tanto tutti parlano, dobbiamo fare questo passo assieme. Dobbiamo poi Dobbiamo poi fare un altro passo dicendo sì alle ulteriori risorse europee sul lavoro, sulla sanità e naturalmente per le imprese. Possiamo anche lasciare perdere le sigle, se a qualcuno non piacciono, ma

Sono risorse necessarie, ma non sufficienti. Ciò che è indispensabile in questo momento è un'unità di intenti qui. Dobbiamo trovare un'unità di direzione in

sconti. Le risorse per la cassa integrazione, per il reddito di cittadinanza, per il reddito di emergenza, per le indennità finiscono, perché sono fondi, in questo momento, a debito e il debito dell'Italia deve restare sostenibile. Ciò che resta da fare, allora, è rimboccarsi le maniche (come si dice da noi al Nord: «*tasi e lavora*»), quindi remare e lavorare, studiare e continuare a remare, facendo fatica per portare la nave Italia fuori dalle secche e possibilmente a veleggiare, magari anche meglio di come abbia fatto da sempre nella storia della Repubblica.

molti colleghi giustamente hanno evidenziato il problema che non è stato possibile per il Senato discutere su un provvedimento così corposo e così importante. Il problema è serio ed è giusto non sottovalutarlo; ragioniamo pure su eventuali modifiche regolamentari, ma io credo - lo voglio dire perché lo penso - che, a partire dal Governo, ci debba essere uno sforzo per organizzare i lavori, insieme alle due Camere, al fine di assicurare il contributo del Parlamento. Per la verità, come anche diversi colleghi dell'opposizione sanno, chi ha tentato di fare, prima in Aula alla Camera, un ragionamento anche con le opposizioni, magari per riuscire a spacchettare questo provvedimento, non è riuscito, né nella maggioranza, né nell'opposizione, a trovare un'intesa. oltre al lavoro sul Regolamento, tutti (Governo, maggioranza e opposizione) dobbiamo provare a trovare - credo sia possibile un modo per organizzare i lavori parlamentari che consenta il contributo del Parlamento. Sarebbe una cosa utile al Governo e più che sacrosanta per le prerogative del Parlamento. Se poi vogliamo essere obiettivi, ormai purtroppo un monocameralismo materiale è in corso da diverso tempo. colleghi: nessuno di noi in quest'Aula può alzare l'indice contro gli altri, perché nel passato ci siamo trovati di fronte (non voglio ricordare l'approvazione del primo bilancio di questa legislatura) a situazioni simili. Se vogliamo provarci, occorre uno sforzo di responsabilità di tutti, *in primis* del Governo e, come direbbe Eduardo, in proporzione: la prima responsabilità del Governo e della maggioranza, ma una responsabilità un'altra considerazione politica da fare. Colleghi, mi è chiarissima la dialettica tra maggioranza e opposizione: ribadisco sempre che è il sale della democrazia. Sento parlare di provvedimento «assistenziale». Ho ascoltato attentamente il dibattito di ieri e di oggi,

una richiesta di ulteriori risorse a pioggia. Lo capisco, perché siamo in questa situazione, ma poi sento poi sento parlare di elezioni e allo stesso tempo ascolto le giuste preoccupazioni - che condivido - in relazione alla situazione economica del Paese.

parlare in questo momento di elezioni. È del tutto legittimo, perché le elezioni sono il punto più alto della democrazia, ma ha

Oppure bisognerebbe fare qualche altra valutazione, decidere che c'è un pezzo di strada che bisogna provare a fare insieme per evitare quei conflitti sociali di cui siamo preoccupati? Infine, altra considerazione e altra domanda: davvero su questi provvedimenti non c'è nulla che vada bene? Davvero possiamo pensare che sia tutto un disastro? È il messaggio giusto che stiamo dando al Paese? Francamente credo di no. Ho ascoltato Bagnai che ci ha

Intendiamoci: noi sul tema della cassa integrazione e sul tema del sostegno alle partite IVA stiamo facendo una cosa che non si è mai fatta in questo Paese. Mai la dimensione della protezione e della tutela ha avuto uno spettro così ampio. È assistenzialismo? Colleghi, non è assistenzialismo; se non avessimo avuto la possibilità di dare la cassa integrazione anche alle imprese sotto i cinque dipendenti e al commercio, se non avessimo aiutato le partite IVA, dove saremmo oggi? Quali sarebbero i dati sull'occupazione? Quale sarebbe la pressione e la crisi sociale?

che c'è uno sforzo enorme e inedito. Questo, colleghi, dovreste riconoscerlo anche voi, non usciremo da questa crisi se non gestendo l'emergenza e costruendo un impianto strategico per questo Paese

delle strumentalizzazioni che troppo spesso pervadono il nostro dibattito. In questo provvedimento ci sono tanti interventi corposi; ne voglio citare due, uno dei

prestiti ha un valore di 286 miliardi di euro: vi sembra qualcosa di poco conto? Risolve tutti i problemi? No. Ma vi sembra qualcosa di poco conto? Insomma, a me piacerebbe che ci fosse la critica, la più aspra, ma che ci fosse anche il riconoscimento di uno sforzo che oggettivamente questo Paese sta facendo

la questione degli affitti (che pure non è risolta). Ci sono interventi importanti - voi dite a pioggia o assistenziali - che cercano di dare una mano a una situazione sociale

un fondo importante per la riqualificazione turistica che possa dare ai nostri operatori una risposta sul futuro e sulla prospettiva, perché, senza questa scelta, limitarsi a rincorrere l'emergenza non ci consentirà di fare un salto di qualità. diamo il nostro voto di fiducia e auspico che con il nuovo scostamento sia possibile affrontare quelle questioni delle quali non è stato possibile occuparci con questo provvedimento. Signor Presidente, sottosegretario Misiani, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che la pandemia ha travolto i saldi di finanza pubblica. Se alziamo per un attimo lo sguardo alle previsioni contenute nella legge di bilancio ci accorgiamo che quei saldi sono ormai un relitto del passato

Non disponevamo - come tutti gli altri Governi in Europa e nel mondo - degli anticorpi per prevenire una pandemia, che è nata *local* e che è via via diventata *global*, in maniera simmetrica in tutti i continenti, ma anche e soprattutto con tempi e modalità che impattano ancora negativamente sui dati macroeconomici. Parlando dell'Italia, un Paese a forte vocazione di *export*, questo rappresenta un'ulteriore insidia alle dinamiche della crescita. Basterebbero, dunque, pochi numeri: i 2.500 miliardi di euro di debito consolidati nel maggio di quest'anno significano che l'Italia sta affrontando una fase molto delicata. Si può ascoltare di tutto, ma siccome non vogliamo partecipare al festival delle banalità, dobbiamo ricordarci che questi numeri ci indicano innanzi tutto che il nostro Paese è tra quelli in Europa che ha utilizzato il maggior tasso di indebitamento, anche rispetto agli altri Paesi europei, per affrontare la pandemia, per proteggere il lavoro e per garantire all'impresa e alle famiglie la liquidità necessaria, per non impedire un futuro migliore alle nostre imprese e alle nostre famiglie. Se prendiamo i dati - se non vi fidate delle relazioni tecniche, neanche di quelle del governatore della Banca d'Italia - ci accorgiamo che l'entità e la percentuale di indebitamento netto che l'Italia ha proposto con le misure per contrastare la pandemia è tra le più alte, insieme alla Germania, di tutta l'Unione europea.

perché dobbiamo tener conto che quando usiamo delle parole pesanti che sono macigno alla credibilità delle istituzioni non svolgiamo una funzione utile agli interessi nazionali. Lo dico con grande franchezza: non sono d'accordo quando ci si accusa di incrinare la democrazia o minacciare che siamo in presenza di una contrapposizione con le regole fondamentali della democrazia. Non credo neanche che sia utile per nessuno definire questo Parlamento «invisibile» perché il Parlamento è il luogo fondamentale dell'attività legislativa e, dunque, è preziosissimo per garantire tutti gli interventi necessari per attraversare la crisi. Noi abbiamo fatto una proposta perché dentro questa emergenza è naturale che i sessanta giorni di tempo per convertire i decreti-legge non siano compatibili con tre letture. Lo abbiamo già visto; è successo in passato, quando non eravamo in emergenze e, a maggior ragione, la decretazione oggi è ancora più compatibile con le caratteristiche dell'emergenza che la Costituzione richiama. Noi abbiamo avanzato una proposta molto semplice, lo dico ai colleghi e approfitto della presenza del Governo. Abbiamo posto solo una condizione di fronte a provvedimenti ampi e complessi: e complessi: spacchettare da subito il provvedimento costruendo un'intesa politica e dividere gli argomenti e i temi tra le due Camere perché solo così si possono rispettare i sessanta giorni che la Costituzione attribuisce.

ma probabilmente non l'ultimo per complessità - richiedano una forte condivisione politica. Colleghi, non è compatibile dividere il Parlamento tra chi lavora e chi no, tra chi conosce il mondo del lavoro e chi no, tra chi porta qui istanze legittime e individuali di disperazione e problematiche che esistono nella popolazione e chi no. Penso a chi come noi ogni giorno vive nella sua quotidianità il rapporto con il mondo del lavoro, con la sofferenza di chi il lavoro lo perde, a chi come noi ogni giorno vive la complessità di realizzare investimenti da parte di coloro che vogliono produrre lavoro, chi, insomma, viene dalla radice del lavoro e del rapporto tra lavoro, impresa e capitale. Insomma, è inaccettabile l'accusa che ci avete rivolto ed è anche poco dignitoso da parte di chi intende difendere il mondo del lavoro portare qui esemplificazioni e letture senza tener conto del contesto complessivo nel quale il mondo e il Paese si sta muovendo per attraversare questa pandemia. Rivendico questa differenza. Probabilmente siamo diversi innanzitutto per questa ragione: noi crediamo che il distanziamento fisico, che è stato necessario per attraversare la pandemia, non debba diventare un distanziamento permanente delle dinamiche sociali. Abbiamo bisogno di ripristinare comunità; noi non mettiamo in contrapposizione la necessaria attività di assistenza, di aiuto e di protezione della popolazione che abbiamo compiuto. Il reddito di emergenza e anche probabilmente un reddito di cittadinanza più orientato a offrire un'opportunità formativa per l'inserimento sono strumenti fondamentali per prevenire conflitto sociale e costruire comunità. Non c'è nessuno spazio per attrarre nuovi investimenti senza garantire coesione. coesione. Quando usiamo le parole, credo dunque sia molto importante dirci tra noi che le scelte che abbiamo compiuto prima nel cura Italia, poi nel decreto-legge liquidità e poi oggi con il decreto rilancio, proprio per garantire un'universalità nella protezione degli ammortizzatori sociali a tutti (cosa mai fatta prima d'ora), un intervento che segna l'identità di questo Governo e le modalità con le quali l'Esecutivo ha inteso attraversare la crisi e affrontare la pandemia. Siamo consapevoli che ci possono essere stati e ci saranno ritardi, che vanno corretti e migliorati, ma basta anche in questo caso un numero. Le ore di cassa integrazione del mese di aprile sono state pari all'intera annualità del 2008, quando la crisi finanziaria che si innestò determinò una complessa crisi economica (le ore di cassa integrazione di un mese sono cioè pari alle ore di cassa integrazione di dodici

Insomma, un conto è denunciare il limite della temporalità dell'erogazione, un altro è mettere in discussione strumenti o accusare questo Governo di incapacità nel dare risposte universali, che invece ha dato proprio al mondo del lavoro. Perché per noi il lavoro, prima di tutto, non è una parola; è un'identità, sulla quale questo Governo ha inteso attraversare la pandemia e superare la crisi. la crisi. Dico con grande franchezza che queste azioni, che sono state importanti e che anche il decreto rilancio ha inserito, sono finalizzate a salvaguardare una questione ancora più grande e più importante. La liquidità delle imprese, infatti, e anche le modalità con le quali noi stiamo attraversando questa crisi generano, insieme agli interventi per le famiglie, una risposta adeguata al nostro Paese, un'identità precisa relativamente a come attraversare la crisi. È per questo che non vogliamo sottovalutare il percorso che è stato costruito. in questa fase le opposizioni, anche ieri, ci hanno parlato di sussidi come di un'attività sbagliata, noi crediamo invece che assistenza, coesione sociale e comunità siano indispensabili per promuovere nuovo sviluppo. Mentre voi parlate di *flat tax*, noi abbiamo prorogato il versamento dei tributi al prossimo 16 settembre, abbiamo soppresso le clausole di salvaguardia dei relativi aumenti dell'IVA e delle accise (misura strutturale utilissima per il nostro bilancio e per il futuro di questo Paese), e abbiamo anche tagliato il saldo e l'acconto IRAP nel 2020 per le imprese fino a 250 milioni di euro di fatturato. E aggiungo che, mentre voi facevate la propaganda sulla *flat noi abbiamo introdotto misure utili a sostenere la liquidità, anche a fondo perduto, delle imprese. E questi sono fatti. Dico, allora, con grande chiarezza ed evidenza che, probabilmente, questo è l'unico Parlamento in Europa nel quale le opposizioni, ogni due per tre, invocano le elezioni. Questo è l'unico luogo, l'unica democrazia occidentale nella quale l'opposizione, in tempo di pandemia, chiama alle elezioni, anziché alla responsabilità istituzionale per attraversare questa fase. Di fronte a noi, abbiamo tre grandi obiettivi sui quali dobbiamo lavorare. Il primo è il nuovo scostamento, necessario per garantire le risorse ai Comuni, indispensabile per finanziare gli ammortizzatori. Abbiamo però di fronte a noi anche l'esigenza di riformare gli ammortizzatori e di salvaguardare quella coesione istituzionale fondamentale tra Stato, Regioni ed enti locali, necessaria per costruire sviluppo economico e crescita. Di fronte a noi, però, abbiamo anche due grandi opportunità: il volto nuovo dell'Europa. Una grande occasione per dare un sviluppo alla *green economy*, alla riduzione del consumo energetico, all'economia circolare, alla riconversione in chiave ecologica dell'economia: significa occupazione, lavoro, crescita. Di fronte a noi abbiamo anche l'occasione fondamentale per un grande, straordinario, piano digitale. Un *new deal* digitale del nostro Paese, altro che il ritorno al contante, come qui è stato evocato come misura fondamentale. Abbiamo bisogno di ridurre le distanze. Ogni chilometro di alta velocità, ogni chilometro di fibra ottica portata nelle nostre abitazioni significa ridurre le distanze, modernizzare questo Paese ed appropriarci, anche con il sistema pubblico, delle nostre più importanti infrastrutture, per costruire crescita e competitività. Questa è la sfida che abbiamo di fronte a noi. Il sovranismo, l'individualismo, l'idea per la quale ciascuno fa da solo per uscire da questa crisi, sono stati sconfitti. Ora tocca a noi costruire una nuova fase economica.

il punto di svolta delle sorti del Paese, ma ci accontenteremo. Oggi, con l'approvazione di questo decreto-legge dal nome così evocativo, si poteva dare avvio a una nuova rinascita; oggi poteva e forse doveva essere una giornata di speranza per gli italiani; oggi doveva essere il giorno del rilancio dell'Italia, del rinascimento del nostro Paese. Avevo immaginato questa giornata senza un voto di fiducia; la immaginavo come la fine di un percorso di condivisione, perché, pur nelle diversità che ci fanno stare agli antipodi di questo emiciclo (e non solo), si poteva seguire un percorso comune per il vero rilancio del nostro Paese. Paese. Infatti, si può anche giocare in squadre diverse, ma sono convinta che se le opposizioni fossero state davvero coinvolte oggi non ci sarebbe stato bisogno di un voto di fiducia, perché se al decreto-legge rilancio in esame avessimo lavorato tutti insieme, se il Governo avesse ascoltato le nostre proposte, oggi noi avremmo davvero reso un buon servizio al Paese, ma purtroppo non è così. Gli italiani avrebbero meritato qualcosa di più che 252 252 pagine e 266 articoli che, come ha scritto testualmente «Il Sole 24 Ore» e non le opposizioni, sono «un'accozzaglia di norme, normette, prebende, violazioni, scorrettezze che reclamano vendetta». pagine vuote destinate a scontrarsi con una realtà molto più dura di quella che raccontate in quest'Aula e al Paese intero. Quello in esame è un ulteriore decreto-legge blindato che il Senato non può fare altro che ratificare, perché non è arrivato in tempo utile per apportare modifiche o miglioramenti. Ci avete servito un piatto cotto e mangiato, senza offrire ai commensali alcuna possibilità di replica. Avete reso il Senato un vero e proprio fantasma. Vi siete riempiti la bocca davanti alle telecamere dicendo che il Parlamento non doveva andare in vacanza. Ebbene, noi siamo rimasti qui, noi qui eravamo; ci avete tenuto ostaggio delle vostre divisioni mentre la gente moriva di virus o di fame e noi impotenti a guardare i vostri disastri. Siete talmente occupati a pensare soltanto alle poltrone da spartirvi che non avete idea di cosa succede fuori da questo palazzo. Basta guardarsi intorno: negozi che chiudono e che non hanno riaperto dopo il *lockdown,* lavoratori che ancora attendono la cassa integrazione come se fosse la manna dal cielo (giustamente ormai è diventata una grazia divina), interi settori che rischiano il collasso; i commercianti sono in ginocchio, i guadagni ancora ridotti non consentono loro di coprire le spese per le forniture, il personale e l'affitto e di certo tutto questo non può essere compensato con un misero *bonus* da 600 euro. Per molti di loro mettere i prodotti in liquidazione e abbassare la saracinesca purtroppo sarà l'unica soluzione. Siete riusciti a dire no anche alla nostra proposta di credito di imposta per pagare gli affitti degli esercizi commerciali, ma vi chiedo: chi non lavora, secondo voi, come diavolo fa a pagare l'affitto? Io veramente ve lo chiedo in modo semplice, sincero. *(Applausi)*. Penso a parrucchieri, estetiste, artigiani, gestori di bar, ristoranti, *pub,* pizzerie e poi ancora a partite IVA, professionisti: sono tutte persone che voi avete tradito con promesse non mantenute. Chiedevano il pane e voi nel frattempo, ubriachi della vostra sete di potere, avete perso il contatto con il mondo reale. I numeri della cassa integrazione, abbiamo sentito, sono impietosi. L'INPS ha lasciato senza assegno quasi un milione di lavoratori che ne avevano diritto e che non hanno ancora visto un euro I fortunati che li hanno visti devono ringraziare gli eroi che in questo Paese non smettono di fare impresa, quelli che il signor Tridico ha il coraggio di chiamare pigri il signor Tridico, quello del *click,* dei numeri della cassa integrazione inventati perché forse preferisce giocarli al lotto, quello del fantomatico attacco *hacker.* La responsabilità, però, non è soltanto di Tridico, perché la responsabilità è del Governo che ancora gli garantisce gli stare seduto su quella poltrona. Vogliamo parlare dell'industria turistica, visto che siamo in estate? Tale industria dà da vivere a oltre quattro milioni di famiglie. Basta guardare le spiagge: sono semivuote, anzi sono praticamente vuote; se n'è accorta anche mia figlia Vittoria di dieci anni. Non vi siete accorti del dramma che sta vivendo questo settore. Non solo non si è decretato lo stato di crisi, come avevamo chiesto noi peraltro, ma siccome siamo nel Paese dove bisogna cantare e bisogna portarsi

situazione di emergenza *(Applausi)*, avete però pensato di regolarizzare gli irregolari. Parliamo di famiglie. Il Governo ha dimostrato di dimenticare totalmente il mondo dell'infanzia. Ci sono madri che hanno rinunciato a tornare a lavoro per accudire i loro figli, perché è mancato il giusto supporto da parte del Governo ai servizi per l'infanzia

un *record* storico. Ma voi pensate che basti mettere due persone nella stessa casa e tenerle in casa chiuse in isolamento forzato per fare figli? Non funziona così, signori cari. Per costruire una famiglia bisogna avere coraggio; per costruire una famiglia serve sicurezza per poter programmare una vita strumenti di conciliazione lavoro-famiglia e non i vostri *bonus* a mo' di mancette che spariranno da un giorno all'altro. Se si parla di figli, non posso non parlare del capitolo rovente della scuola. Sul nuovo anno scolastico è andato in scena il teatrino dell'assurdo, tra *plexiglass*, *software* per misure dei banchi ergonomici e delle dimensioni delle aule. Insomma, milioni di studenti che ancora non sanno dove andranno a sedersi perché la Azzolina ha detto che un milione di bambini deve stare fuori, stare fuori, forse al parco, forse sotto un fico come ai tempi di Socrate probabilmente. In quest'Aula abbiamo chiesto tutti, dalla Lega, a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, le dimissioni del ministro Azzolina. per dimettersi, anche se si è stati commissariati (perché questo è successo), serve dignità e probabilmente la parola «dignità» la sapete scrivere soltanto su decreti che poi diventano inutili. Siccome sappiamo che c'è il blocco dei licenziamenti, facciamo un'eccezione alla regola e licenziamo la Azzolina. Ecco, questa è la l'unico caso in cui probabilmente anche i sindacati farebbero una *ola* e non solo gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e tutto il personale. E veniamo ai *reality* ai quali vi ispirate, ai vostri cavalli di battaglia, parole usate ed abusate per ingannare gli italiani. «Fondo perduto»: questo sconosciuto; portatemi qui dieci persone che hanno preso i soldi a fondo perduto, perché io sono sfortunata e non ne ho incontrata neanche una. Poi, «garanzie»: 400 miliardi di euro dei quali agli sportelli bancari - che forse non conoscete - sono rimasti soltanto la frustrazione di chi fa ore di coda ogni giorno per poi non ricevere nulla. Sul fronte fiscale, aziende e professionisti non sono considerati risorse per dare benzina all'economia, ma veri e propri bancomat da spremere. giorni ci saranno 246 scadenze fiscali: tutti versamenti, ossia tasse da pagare. Noi chiedevamo un anno fiscale bianco, ma nemmeno il minimo sindacale è stato fatto. Il rinvio di adempimenti fiscali al prossimo autunno i commercialisti lo hanno chiesto questa mattina su molti quotidiani affermando che «il buon senso lo impone». Peccato che ci siamo resi conto che questo Governo è contro il buon senso: questa è la verità. Avete annunciato un altro scostamento di bilancio. Prima diteci dove sono andati a finire i soldi e come sono stati spesi gli 80 miliardi di euro di due scostamenti di bilancio per le cui approvazioni i voti dell'opposizione sono stati fondamentali. Noi, questa volta, di voi non ci fidiamo. Quindi, prima vedere cammello e poi votare scostamento, perché non indebiteremo più i nostri figli e i nostri nipoti al solo scopo di garantirvi la permanenza al Governo. In conclusione, il provvedimento in esame è solamente uno dei tanti disastri di questo Governo, che distrugge tutto quello che tocca. Noi però non ci renderemo mai complici della distruzione dell'Italia. C'è un detto che dice che chi non conosce i propri limiti ha il destino segnato. Bene, di voi non si occuperà la storia:

E così sarete relegati nel girone degli ignavi. Noi siamo dalla parte di chi oggi soffre ed è stato illuso. Per questo motivo, Forza Italia dice no al provvedimento in esame e voterà no alla fiducia. Siamo e resteremo sempre all'opposizione del Governo Conte, che si è dimostrato incapace di gestire tutti i *dossier* finora osservati e inadeguato ad affrontare le sfide che l'Italia si è trovata di fronte. Fatevene una ragione.

il Governo rinvia le decisioni a decreti attuativi che sono tutti da costruire e realizzare e che potrebbero non vedere mai la luce. Di fronte a questa situazione, in cui il Parlamento di fatto non ha più poteri, abbiamo assistito negli ultimi mesi a continui interventi della maggioranza in cui si accusa noi - la minoranza di centro-destra e la Lega - di non avere un atteggiamento responsabile. Noi rimandiamo al mittente quest'accusa, perché abbiamo dimostrato di a favore di quei provvedimenti utili al Paese. Mi riferisco allo scostamento di bilancio. È stato ricordato dal Capogruppo, senatore Romeo, che noi siamo stati determinanti per lo stanziamento di quei 55 miliardi di euro che voi oggi volete spendere in questo modo così dissennato.

Vedete, questi dibattiti assomigliano spesso a un teatro dove ognuno interpreta una parte, ma, a differenza del teatro, c'è un giudice che poi, alla fine, decide chi aveva ragione e chi torto, chi ha interpretato correttamente le esigenze del Paese e chi invece non l'ha saputo fare. E quel giudice è il popolo. *(Applausi)*. Nelle vostre invettive potete dissertare di quello che volete, ma il popolo si esprimerà prima o poi; potete rinviare all'infinito le elezioni, ma prima o poi quel giorno arriverà. Vi ricordo che la Lega, come forza di Governo, in un anno è passata dal 17 al 34 Voi avete dimezzato i vostri consensi dimostrando di non essere in sintonia con il Paese e all'altezza di governare l'Italia, passando dal 32 al 17 Questi sono i fatti, al di là delle chiacchiere che possiamo fare, da destra a sinistra, sulla coerenza e sull'attività di maggioranza e opposizione. Noi continueremo con il nostro atteggiamento responsabile,

decreto liquidità è stata una presa in giro, con il famoso *bazooka* dei 400 miliardi, che non ha messo un euro in più nelle tasche della maggior parte dei cittadini e delle aziende italiane. Ora, il decreto rilancio rappresenta un'occasione persa. Abbiamo

eccezionale, autorizzata dall'Europa per l'emergenza Covid e per certi versi irripetibile, tanto da determinare che questi soldi dovessero essere spesi bene, occasione che non doveva essere persa. È questo che vi contestiamo. C'erano di fatto due modelli per spendere queste risorse: il vostro, quello solito dei *bonus*, dei sussidi e dell'assistenzialismo; e quello che rappresenta invece la proposta della Lega e di tutto il centrodestra, ossia la riduzione della pressione fiscale. Raccogliete soldi in modo spropositato da famiglie e imprese, per poi redistribuirli; noi invece li vogliamo lasciare nelle tasche dei cittadini e delle imprese, perché possano fare investimenti: questo è l'unico modo per renderle competitive, non certamente il prelievo indiscriminato e dissennato che mette fuori mercato le nostre aziende. Grazie a queste politiche, siete i responsabili del declino della nostra economia e del nostro Paese. Questa era Questa era l'occasione da cogliere: non l'avete colta, ma a settembre, quando molte aziende non riapriranno, lasciando a casa migliaia di lavoratori (perché questo è il rischio reale che stiamo vivendo), e finiranno le risorse stanziate e - ahimè - non ancora distribuite della cassa integrazione, risposte darete al Paese? Dopo aver speso questi 55 miliardi, cosa rimarrà delle prospettive di crescita del Paese e delle possibilità di mantenersi per i cittadini italiani? Veramente pensate che questo decreto-legge possa promuovere il rilancio del Paese e della sua agricoltura, ad esempio, con una sanatoria indiscriminata per gli immigrati? È questa la risposta per l'agricoltura che avete messo in campo? Pensate veramente che avrà efficacia e che il settore più colpito, il turismo, che dava al Paese il 13 per cento del PIL e impegnava più di 4 milioni di lavoratori, possa risollevarsi con il *bonus* vacanze, che graverà poi sulle aziende turistiche? Pensate veramente che estendere lo stato d'emergenza fino a ottobre - o peggio, a dicembre - non avrà alcun effetto sulla sensazione di pericolo che avranno gli stranieri nel decidere se venire in vacanza nel nostro Paese È più importante la sicurezza del presidente Conte rispetto alla possibilità di sviluppare il turismo nel nostro Paese? Siete irresponsabili, se lo pensate. Pensate veramente che nel campo dei trasporti, con un settore dell'automobile in ginocchio, tutto si possa risolvere con il *bonus* per l'acquisto di monopattini, fra l'altro neanche prodotti in Italia, senza dare lavoro agli italiani,

Il Gruppo Lega-Salvini Premier non voterà certamente a favore della fiducia a questo Governo. Continueremo a cercare di dare il nostro contributo, come abbiamo sempre fatto, con tutti i decreti che avete posto alla nostra attenzione in questi mesi, e vogliamo farlo fino in fondo, perché torneremo al Governo e abbiamo già le proposte e le idee chiare su come governare questo Paese. Continuiamo a ripeterlo e a ripresentare le nostre proposte e i nostri emendamenti.

ai provvedimenti che stanziano risorse per il nostro Paese; mettetevi bene in testa, però, che non saremo mai complici delle vostre follie, dei vostri errori, delle vostre occasioni perse e delle vostre scelte sbagliate. La Lega non ha fiducia in voi, come la maggior parte dei cittadini italiani, e lo sapete: potete chiudervi in questo palazzo, chiudere le porte, arroccarvi qui dentro e perdere il senso della realtà, come ormai avete fatto da mesi; fuori però c'è una realtà ormai arrabbiata, che non può ancora manifestare fino in fondo il proprio dissenso, e ci sarà purtroppo - sottolineo purtroppo - un autunno caldo, di fronte al quale ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità. Noi dall'opposizione lo facciamo come forza di Governo, perché sappiamo di essere maggioranza nel Paese; voi siete assolutamente inadeguati e le vostre invettive nei confronti dell'opposizione non produrranno niente. Sono parole vuote, che pronunciate in quest'Aula, ma che non trovano nessuna eco all'esterno di questo palazzo. Vi illudete che con le accuse all'opposizione ritornerete ad avere consenso, ma quel consenso che avete perso certamente non lo ritroverete attraverso questo atteggiamento e provvedimenti sbagliati che non risolveranno le sorti dell'economia del nostro Paese. La Lega-Salvini Premier voterà no alla fiducia a questo Governo e a questo provvedimento, che è un'occasione persa per tutti e per l'intero Paese. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a licenziare oggi qui in Senato è uno dei più ingenti e anche dei più criticati e poderosi della storia italiana. Per sostenere imprese, famiglie e lavoratori abbiamo stanziato 55 miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere ai 25 del cura Italia. È il terzo dei decreti economici varati da questo Governo in risposta alla pandemia Covid-19. I tre decreti infatti (il cura Italia del 17 marzo, il liquidità dell'8 aprile e ora il decreto rilancio, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 19 maggio, perché anche la scansione temporale ha la sua importanza), vanno letti come un *continuum* e fanno parte di un unico disegno organico. Con il cura Italia infatti si è inteso dare risposta immediata all'emergenza, che da sanitaria rischiava di diventare economica, potenziando il sistema sanitario, offrendo sostegno al reddito, bloccando i licenziamenti, estendendo la cassa integrazione in deroga, sospendendo la scadenza delle imposte, fornendo risorse alle imprese in difficoltà, avviando finalmente il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e della scuola italiana atteso da anni. Con il decreto liquidità, poi, si sono rese operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, fornendo gli strumenti per l'accesso al credito e alle agevolazioni di diversa natura messe in campo. Ora, con il decreto non a caso chiamato rilancio, si progetta il futuro. Con questo provvedimento infatti non solo potenziano le misure precedenti e proroghiamo i termini delle agevolazioni e degli aiuti previsti, ma disegniamo appunto il futuro del Paese. Non giochiamo quindi solo in difesa, come pure è stato detto, rispetto a un evento imprevisto e drammatico quale la pandemia che si è abbattuta sull'intero globo, ma offriamo una prospettiva di lunga durata per lanciare l'Italia nel futuro. Proprio questo significa infatti l'aver introdotto il super *bonus* al 110 per cento per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico, con in più la possibilità di utilizzare il credito maturato, cedendolo a terzi o alle banche: un'autentica rivoluzione *green*, che non solo consentirà al nostro Paese di migliorare le proprie prestazioni energetiche e rinnovare il patrimonio edilizio, con un risparmio energetico che avrà ottime ricadute sul piano ambientale, che avrà un impatto positivo anche sul mondo del lavoro e agevolerà la creazione di un circolo economico virtuoso, attraverso appunto la cessione del credito. Tale rivoluzione *green* avrà il suo seguito naturale con un ulteriore provvedimento in arrivo, dedicato alla semplificazione e alla sburocratizzazione in materia di contratti pubblici e di edilizia. Nulla è stato dunque lasciato al caso. Da marzo ad oggi, dal momento in cui l'Italia è stata colpita da questa sventura che ha cambiato le nostre abitudini di vita, questo Governo, il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno subito compreso che dalla crisi poteva e doveva nascere l'opportunità di guardare oltre di introdurre finalmente quei profondi cambiamenti che il Paese aspetta da decenni. Uno fra tutti è il potenziamento del Sistema sanitario nazionale e il rafforzamento del sistema scolastico, dal punto di vista sia edilizio sia didattico. Questa emergenza ha reso finalmente chiaro a tutti

si erano stanziate tante risorse per la sanità e per la scuola. Un quadro omogeneo dunque, coerente e lungimirante: ma in quale contesto è stato concepito? Vorrei

che, dopo una sola legislatura all'opposizione, è passata al governo del Paese. Ripercorriamo brevemente, dunque, la storia di questa legislatura che sta giungendo a metà percorso, anche per dare il contesto di riferimento in cui i suddetti provvedimenti nascono. Dopo un travaglio di un paio di mesi, a giugno 2018, si forma il Governo giallo-verde; passano neanche due mesi e ad agosto la tragedia: il ponte Morandi viene giù come una lastra di cioccolato al sole, causando 43 vittime e lo sbigottimento di un Paese intero. Passa un anno e nell'agosto successivo il senatore Salvini decide di fare strame del contratto di Governo sottoscritto e provare a passare all'incasso. Il collega Tosato ha appena simpaticamente ricordato come in quell'anno di governo con noi, la Lega sia passata dal 17 al 34 per cento. Bella forza! Invece di lavorare, avete passato il tempo a fare propaganda. Dell'anno di governo della Lega si ricordano due cose: i decreti sicurezza; in realtà avevano fatto anche il decreto concretezza, ma nessuno sa cosa sia. In ogni caso, il tentativo di passare all'incasso fallisce. Evitiamo il testacoda e si forma il nuovo Governo, quello attuale. Persino sul suo cavallo di battaglia, il contrasto all'immigrazione clandestina, questo Governo sta facendo meglio di lui. La ministra Lamorgese, lontana dai riflettori, dai clamori mediatici e dai *selfie* - 500 Senatrice Marin, si segga, per cortesia! MAIORINO *(M5S)*. La ministra Lamorgese, lontana dai riflettori e dai clamori mediatici, ha decuplicato il numero dei ricollocamenti

Dopo pochi mesi dalla formazione di questo Governo, ecco abbattersi sull'Italia e sul globo intero niente di meno che una pandemia. Questo è stato il percorso a dir poco accidentato che abbiamo attraversato e che ci ha condotto fino ad oggi, al voto su questo decreto rilancio: oggi, quel 14 agosto 2018 torna prepotentemente attuale. Io, come penso tutti voi in quest'Aula, ricordo molto bene quel giorno. Rimasi con il fiato sospeso per qualche ora, in attesa di sapere

Poi, finalmente, le parole del ministro e collega Toninelli: chiarissime, nette e ineccepibili; le uniche che i genovesi e gli italiani volevano sentire. «Un Paese civile e moderno come l'Italia» disse «non può permettersi di vedere fatti tragici come questo. Non è accettabile. Chi ha sbagliato deve pagare fino alla fine». *(Applausi)*. la prima cosa che faremo sarà guardare la concessione stipulata con Autostrade per l'Italia, revocarla e sanzionare pesantemente coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di manutenzione. Che sollievo furono queste parole, non ce n'erano altre che il mio MoVimento potesse pronunciare in quel momento. Era la reazione giusta, l'unica possibile di fronte a quel disastro. Oggi, finalmente, quelle parole hanno trovato un seguito e una concretizzazione, dopo il durissimo negoziato conclusosi l'altro giorno. La famiglia Benetton sarà estromessa dalla gestione delle Autostrade. Rinuncia ai 23 miliardi di mancato guadagno, cede la partecipazione in Aspi e quindi la gestione dell'infrastruttura. Autostrade per l'Italia diventa una *public company* aperta a nuovi investitori istituzionali e corrisponderà un risarcimento di 3,4 miliardi, rinunciando ad ogni causa contro il conducente, ossia lo Stato. Il piano tariffario dei pedaggi sarà quindi rivisto secondo le nuove indicazioni dell'autorità regolatoria. Ci sono voluti due anni, ma questo passaggio rappresenta davvero il tramonto di un'epoca, in cui per troppo tempo lo Stato aveva favorito pochi piccoli potentati, a danno dei cittadini e dei contribuenti, ossia di quella collettività che invece rappresenta. Ci sono voluti due anni e, come ho ricordato, non sono stati semplici, anzi, piuttosto movimentati. A grandissime linee. questo è il quadro in cui ci siamo trovati ad operare, con un'opposizione che, come abbiamo già denunciato da tempo in quest'Aula, nemmeno di fronte a una tale emergenza ha ritenuto opportuno essere costruttiva e responsabile e pezzi di maggioranza che, non ce lo nascondiamo, talvolta, anziché favorire la collaborazione, sembrano divertirsi a gettare sabbia negli ingranaggi.

Bisogna dire però che i dati sono tali e, al netto di fisiologiche difficoltà, ad oggi abbiamo 850.000 domande di prestito garantito dallo Stato accolte dall'Agenzia delle entrate, per 51 miliardi di euro di finanziamenti erogati. La stessa Agenzia delle entrate ha erogato 4,5 miliardi di contributi a fondo perduto verso 1,4 milioni di piccole imprese. L'INPS, che nel 2009, anno della crisi finanziaria, aveva lavorato e autorizzato 916 milioni di ore di cassa integrazione per tutto l'anno, nella sola metà del 2020 ne ha autorizzate 2 miliardi. Qualcosa si è inceppato? C'è qualche ritardo? Certamente sì, ma il 7 luglio l'INPS ha pagato 7,3 milioni di prestazioni di cassa integrazione, a fronte dei 7,6 autorizzati. Abbiamo cercato di pensare veramente a tutto e a tutti. Concludo dicendo che domani è un giorno cruciale: avrà avvio un Consiglio europeo straordinario, che molto probabilmente stabilirà i destini dell'Italia e della stessa Unione europea. Sappiamo bene che non sarà un passaggio semplice. È notizia di oggi che alcuni Paesi si oppongono fieramente alle proposte portate avanti dall'Italia e supportate anche da Francia e Germania. Ribadiamo dunque la nostra fiducia nel presidente Conte, certi che saprà mettere a frutto il grande lavoro svolto negli scorsi mesi: a lui vanno il nostro sostegno *(Applausi)* e la nostra fiducia e a questo Governo annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle. nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni,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

Arrigoni).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello. Ho un elenco di 17 senatori che hanno chiesto di votare

Cesaro,

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo,

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

il valore di tutta l'operazione è aumentato in modo esponenziale. L'altro elemento assolutamente allarmante riguarda la relazione governativa annuale sull'*export* di armamenti, che è stata trasmessa al Parlamento proprio nel mese di maggio

Vorrei ricordare che la legge 9 luglio 1990, n. 185, regola la vendita all'estero dei sistemi militari italiani, vieta espressamente le esportazioni di armamenti verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani aggiungendo anche che che le esportazioni devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e anche all'articolo 11 della Costituzione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, rispondo al quesito della presidente De Petris sulla base degli elementi forniti dal Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, impossibilitato a partecipare alla seduta. Le decisioni sulle forniture nel settore della difesa comportano due ordini di valutazioni, entrambi importanti: un controllo tecnico e un vaglio politico. Sulla base della legge n. 185 del 1990 il Governo esamina caso per caso le richieste delle imprese italiane di autorizzazione a trattative contrattuali. In un secondo momento, se le trattative hanno portato alla firma di un contratto, valuta l'autorizzazione all'esportazione. Il Governo esamina la specifica natura delle forniture, il destinatario, l'utilizzatore, la loro possibile destinazione d'uso. Gli accertamenti vengono effettuati anche attraverso il contributo di pareri tecnico-militari.

in materia di diritti umani. Le violazioni devono essere accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dall'Unione europea o dal Consiglio d'Europa. Per quanto riguarda nello specifico le fregate Fremm, il Governo ha effettuato un'attenta disamina sotto il profilo tecnico giuridico a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla deliberazione dell'Unione europea. Naturalmente ha valutato anche gli aspetti prettamente politici della questione. Sotto questo aspetto va tenuto in considerazione il ruolo svolto dall'Egitto nel Mediterraneo allargato, dalla lotta al terrorismo e al contrasto del traffico di esseri umani, dalla tutela dei nostri interessi energetici alla crisi libica. Questo vaglio è oggetto di una successiva e distinta procedura di valutazione che, nel caso specifico, è in corso. Tengo a precisare che nessun altro Stato europeo ha finora adottato misure restrittive su questo tipo di materiali, mancando del tutto un riferimento ad eventuali violazioni nelle attività di ordine pubblico interno. Tali valutazioni e scelte non incidono minimamente sulla nostra ferma e incessante ricerca della verità sul barbaro assassinio di Giulio. La sua tragica morte è una ferita aperta per tutto il Paese. La richiesta di giustizia rimane profondamente radicata nell'opinione pubblica, in questo Parlamento e in tutte le istituzioni, Governo in prima fila. Non cesseremo di esigere ad ogni occasione la verità. Per tutti noi è un impegno ben chiaro, una responsabilità che sentiamo forte nelle nostre coscienze.

per una vendita di armi molto consistente. La violazione dei diritti umani non è un fatto o una questione di ordine pubblico all'interno di un Paese. La vicenda dell'Egitto, come Amnesty international

che non si chiuda la questione delle vendite ed, anzi, che ci possa essere un'operazione che sarebbe molto importante per il prestigio del nostro Paese, che significherebbe anteporre innanzitutto il rispetto dei nostri cittadini e i diritti umani a qualsiasi tipo di affare.

media. I media sono concentrati su tali questioni, sull'utilizzo della Cassa depositi e prestiti e sulla difesa del risparmio postale, oltre che naturalmente su quello che è l'investimento, e qui si tratta veramente di un investimento. Questo risultato è frutto di un'operazione confusa e un po' violenta. Noi le chiediamo di vederla oltre che nella parte societaria, prettamente finanziaria, che probabilmente ha competenze di altra delega, nella linea politica perché il Governo è un organo collegiale. Le chiediamo però di vederla anche rispetto alla sua delega di Ministro per le partecipazioni statali e, quindi, di gestore della politica economico-produttiva e industriale del nostro Paese. Certo, chi le parla vorrebbe che lo Stato non facesse l'imprenditore e si occupasse di scuole, ospedali, giustizia e difesa; governa lei e io mi oppongo. Ma le chiediamo: qual è il riflesso industriale e occupazionale di una scelta di questo genere? Quali le conseguenze, anche sul gruppo Benetton, rispetto al marchio tessile e alla sua presenza nel mondo? Molte delle aziende presenti sui tavoli di crisi, che citiamo nell'interrogazione, hanno soci esteri. la situazione? Si fideranno ancora? Si fideranno dell'Italia e degli impegni che dovrà assumere su quei tavoli, in alcuni casi, per uscire dalla crisi? Si parla di abbassare le tariffe

Non pensa che questo modo di agire acutizzi uno scontro tra Stato e imprese? Abbiamo bisogno di pace. Abbiamo bisogno di sicurezza.

Rispondo - perché correttamente la domanda è posta in questi termini - dal punto di vista industriale. Io credo che in uno Stato liberale come il nostro, in un'economia liberale come la nostra, sia lo Stato a fare regole, lasciando che gli imprenditori giochino sul tavolo delle regole, certe e uguali per tutti. Questo è l'obiettivo che questo Governo ha. Ciò considerato, siamo in un momento di grande complessità, come è evidente, dal punto di vista economico e industriale.

deve essere una guida importante, anche attraverso le grandi aziende partecipate dallo Stato. Come molti sanno, le grandi partecipate sono a disposizione non

di Terna, ad esempio per la parte elettrica, di Snam, per la parte gas, di ENI, per la parte *oil & gas*, e di Leonardo, per altri *asset* importanti della nostra economia. La parte di infrastrutture materiali come quella autostradale è un *asset* strategico e importante; può essere un vantaggio per lo Stato essere presente, soprattutto perché quello non è un mercato concorrenziale.

Credo, quindi, che possa essere un *asset* importante, in cui lo Stato può rappresentare una guida; certamente avrà alcune capacità, che sono quelle di guidare meglio le necessarie manutenzioni e implementazioni dei nostri sistemi di trasporto. di un'operazione fondamentale per il nostro Paese. Altrettanto sarà fondamentale la presenza dello Stato nella gestione della rete unica per la digitalizzazione del Paese; in parte c'è già, attraverso Open Fiber, di cui Cassa depositi e prestiti è già, assieme ad Enel, azionista di riferimento. Credo che in questo momento storico sia necessario che lo Stato investa in alcune infrastrutture: quella autostradale è una di quelle, a nostro avviso, fondamentali. al di là di tutti gli altri punti di vista, sotto i quali si può vedere il *dossier* ASPI, credo che dal punto di vista industriale sia proprio giusto e intelligente per lo Stato investire.

avviso rischia di creare sfiducia in Italia, dichiarando la nascita di un nuovo sistema di partecipazione statale, dopo aver faticato tanto a smantellarlo ed evitando di metterci i soldi degli italiani. Noi abbiamo il grande timore che faccia fuggire dall'Italia molti investitori per le modalità con cui è stata avviata, non tanto per la gestione che valuteremo. Gli investimenti in Italia - lei sa bene

continua a dichiarare la revoca eventuale delle concessioni. Finisco sulla questione Benetton, ma che vada a verbale: non compete a lei l'azione, ma l'ipercomunicazione

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche se in ambito europeo l'attenzione è sempre polarizzata dalla contrapposizione rigore *versus* flessibilità, non c'è dubbio che la questione legata alla difesa e alla sicurezza sia uno dei punti più delicati dell'agenda dell'Unione europea. Il dato positivo è che in questi ultimi anni abbiamo assistito a una netta accelerazione dell'integrazione della difesa europea. Su altri temi il progetto europeo ha difficoltà a darsi dei correttivi, mentre diversi fattori,

che nel contesto di oggi riguarda l'autonomia strategica dell'Unione come attore nello scenario geopolitico internazionale e nella competizione economica e tecnologica globale. Ovviamente l'Italia è il centro di questa dinamica, perché è al centro dell'area del Mediterraneo, uno dei fulcri mondiali di instabilità. Inoltre, perché è Paese a forte vocazione europeista e perché abbiamo un sistema industriale di primo livello di eccellenza assoluta. In tale quadro hanno una funzione essenziale i programmi destinati ad essere finanziati nell'ambito del Fondo europeo della difesa nel quadro del bilancio pluriennale europeo di prossimo Per quanto riguarda la cooperazione strutturata permanente, su un totale di quarantasei progetti l'Italia è capofila in nove progetti e partecipa ad altri sedici: si tratta di progetti strategici, tra i quali ha una valenza particolare quello del sostegno militare in caso di catastrofi, emergenze civili e pandemie. Secondo il meccanismo Pesco e Fondo europeo di difesa (EDF) i programmi sono improntati al principio del cofinanziamento e richiedono dunque *pro* quota un adeguato impegno finanziario da parte dei Paesi partecipanti. Una prima fase del progetto va finanziata dai bilanci nazionali, per una seconda una seconda fase arriva il finanziamento UE. Questo vale soprattutto per i Paesi capofila. Per mantenere il ruolo di *leadership* acquisito è dunque necessario stanziare una determinata quota di risorse, altrimenti si rischia di perdere il controllo, il ruolo di capofila o addirittura di essere estromessi dal progetto. La domanda che le poniamo è dunque quali strumenti o procedure possiamo definire per assicurare risorse finanziarie e stabili a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea.

In questo senso, le iniziative per il consolidamento della sicurezza comune, così come i correlati programmi di sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale della difesa, rappresentano un'opportunità che come Paese vogliamo favorire e siamo impegnati a cogliere al massimo grado. Le attuali contingenze economiche e sanitarie e gli sviluppi del contesto geopolitico nelle aree di interesse confermano - semmai ce ne fosse bisogno - che è quanto mai urgente la realizzazione condivisa di un ambizioso sistema di gestione comunitaria, da sviluppare anche ricorrendo a tutte le possibilità offerte dalle iniziative già operanti, a partire dalla Pesco. Al riguardo, la prevista revisione entro l'anno in corso delle sue regole di gestione deve consentire di ottimizzare i progetti di cooperazione, razionalizzandoli anche facendo ricorso alle procedure e ai finanziamenti previsti nel quadro del Fondo europeo per la difesa. Quest'ultimo è infatti fondamentale per finanziare e favorire i programmi cooperativi di ricerca e sviluppo capacitivo in ambito difesa, nell'ottica di poter efficacemente fronteggiare la crisi e le minacce future. Sosteniamo da tempo la necessità di un bilancio ambizioso e adeguato del suddetto fondo, che nel dimensionamento attuale non è ancora sufficiente, con il quale contribuire a sostenere l'economia nazionale ed europea, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Per l'Italia questo significa favorire il comparto produttivo della difesa, da supportare anche con opportuni strumenti di incentivazione finanziaria, considerato il fatto che esso rappresenta un fondamentale settore per la ripresa economica dell'intero Paese. In tale quadro, per quanto attiene specificamente ai programmi di sostegno all'industria della difesa, previsti nell'arco temporale 2017-2020 - la vera e propria prova sul campo di quanto avverrà nel futuro - rappresento che lo scorso giugno la Commissione europea ha ufficializzato il risultato dell'aggiudicazione dei finanziamenti in ambito Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e Azione preparatoria per la ricerca (PADR) per il 2019. Delle 40 proposte industriali presentate in ambito EDIDP, 16 sono state selezionate per il finanziamento, e tra queste due sono a guida nazionale, mentre sette vedono comunque la partecipazione di imprese italiane nel consorzio vincitore. In ambito PADR, in attesa dell'ufficializzazione dell'aggiudicazione 2019, su 18 progetti selezionati, 12 sono a partecipazione italiana, di cui tre in posizione di coordinatore del consorzio. Al fine di definire il volume esatto dei finanziamenti di cui potrà beneficiare l'industria nazionale, sarà necessario attendere la conclusione degli accordi di sovvenzione, dai quali sarà possibile acquisire le definitive quote di ripartizione del lavoro nell'ambito di ciascun consorzio industriale. Ciò anche al fine di poter definire in modo congruo - secondo il principio dell'equo ritorno - la percentuale di contribuzione nazionale a cofinanziamento governativo del progetto in questione. Dai dati attualmente disponibili, e nelle more della firma dei suddetti accordi, è verosimile desumere che, a fronte di circa 200 milioni di euro assegnati dalla Commissione, i progetti che vedono la partecipazione di industrie nazionali in ambito EDIDP saranno beneficiari di poco più di 134 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti circa 12 milioni provenienti dalle progettualità selezionate in ambito PADR. In conclusione, queste cifre cifre devono essere lette in una sola prospettiva: un progressivo accesso del comparto industriale della difesa ai flussi di finanziamento europei, con inconfutabili ricadute sia nell'ambito occupazionale sia in quello del *know-how* tecnologico.

e mantenerlo e renderlo più efficiente sicuramente rappresenta una delle priorità per il nostro Paese, anzitutto sul fronte interno (lo abbiamo visto anche nella gestione sanitaria di questo periodo). tempo, nella prospettiva europeista, che è un argomento sullo sfondo dell'interrogazione, come ha citato bene lei, signor Ministro, la difesa è certamente un tema promettente, anche in un'ottica di di maggiore integrazione europea. La cooperazione europea, anche in ambito industriale, senza dubbio massimizza la spesa e consente un'economia di scala anche per quanto riguarda questo tema. Come diceva bene lei, l'essere riusciti ad aggiudicarsi la *leadership* di importanti progetti europei è un segno di vitalità e di eccellenza per il comparto industriale del nostro Paese. Sono progetti essenziali per la capacità europea e sostengono un settore industriale importante che ha avuto una contrazione in questo periodo.

*(FdI)*. Signor Ministro, facendo la premessa che i dati sul Covid, come avrà avuto modo di vedere, nelle ultime settimane sono assolutamente confortanti e aggiungo: grazie a Dio. infatti, ormai 57 pazienti in terapia intensiva e i nuovi contagi a ieri erano 162. Abbiamo visto che parte della scienza che sicuramente si è divisa - sostiene che questo maledetto virus è clinicamente morto. Cito il professor Zangrillo per nominarne uno. uno. Mi fido moltissimo dei clinici perché sono medici che sono stati e continuano a stare in trincea, che stanno al fianco dei malati e che hanno potuto vedere esattamente qual era la situazione.

che molti uccelli del malaugurio ci dissero che i contagi avrebbero avuto un'impennata; hanno usato appellativi come delinquenti, disgraziati e irresponsabili. questo caso, grazie a Dio, tutto ciò non è successo, tant'è che il Governo ha cominciato a fare delle riaperture: si sono aperti cinema, teatri, concerti di musica lirica, ristoranti e discoteche all'aperto.

al chiuso e, quindi, non riusciamo a capire quali siano le motivazioni che continuano a perdurare in questa situazione di stallo. Lei, essendo il Ministro dello sport, sa bene il prezzo altissimo che ha pagato il calcio con con la sospensione di tutti i campionati. Al di là della partita in sé, lei sa che ci sono milioni di italiani che hanno passione e vi trovano svago. In un momento così drammatico, sicuramente sarebbe stato un aiuto. Le chiedo, allora, di accogliere le richieste delle federazioni sportive e dei e dei tifosi - anche il collega, senatore La Russa, più volte in quest'Aula ha parlato del tema - per adottare in tempi rapidi delle soluzioni adeguate a garantire un'apertura graduale Le faccio un esempio: io sono di Milano e lo stadio San Siro ha 80.000 posti. Io credo che un terzo degli spettatori potrebbe da subito andare a vedere le partite. Certo, bisognerà tenere conto della specificità degli impianti, della capienza e anche delle squadre e, quindi, le poniamo questo quesito perché vorremmo ridare quella passione e quell'emozione agli italiani che trovano lì un'emotività importante nella loro vita.

poi con gli allenamenti degli sport di squadra e poi finalmente riprendere le competizioni sportive, cosa alla quale - come può immaginare - anche io, come Ministro dello sport e come cittadino italiano, ero particolarmente interessato perché condivido in maniera piena l'idea, di

si ritiene di dover continuare, in qualche modo, proprio su quella linea di prudenza che ci ha consentito, gradualmente, di riaprire le varie attività sportive e semmai prepararci, in maniera perché a settembre, alla riapertura del campionato, che poi significa solamente tra due mesi, ci siano tutte le condizioni per poter riaprire gli stadi e consentire a decine di migliaia di tifosi di assistere alle competizioni sportive. Oggi, se è vero che, all'interno degli stadi, ci sarebbero le condizioni e gli spazi per garantire un distanziamento tra un *tot* numero di tifosi, è anche vero che viene considerato molto rischioso favorire l'afflusso di un numero enorme di persone (ad esempio, appunto, le 10.000-12.000 alle quali lei faceva riferimento nel caso specifico di Milano) che vadano a dirigersi tutte, contemporaneamente, verso un unico luogo, prendendo mezzi autonomi o mezzi di trasporto pubblici. Soprattutto, capire come gestire questo flusso di persone per l'ingresso all'interno degli stadi, con la necessità di misurare la temperatura e fare tutta una serie di che, probabilmente, mancando ormai poco più di due settimane alla fine del campionato (il 2 di agosto), anche insieme alla Federazione e alle leghe, sarebbe difficile organizzare. Il mio impegno, da questo punto di vista molto preciso, è quello, invece, di creare tutte le condizioni affinché quell'auspicio che viene richiamato dalla senatrice interrogante e che io, nello spirito e nell'effetto che produce, condivido pienamente, possa essere attuato a partire dalla ripresa del nuovo campionato nel prossimo mese di settembre.

vita. Vogliamo tornare alla vita di tutti i giorni. Per carità, dobbiamo assolutamente garantire la sicurezza e la salute, ma, dal momento

comportamento sia figlio di una cultura *radical chic* che penalizza gli sport popolari come il calcio. Se lei dice che si può andare a un concerto di musica lirica, se lei dice di sì ai cinema e ai teatri, dove si sta al chiuso, io ho veramente questo sospetto: che non stiate con il popolo, che non stiate con le passioni, che non stiate con gli uomini e con le donne che vi chiedono di smetterla con questa politica del terrore e di farci tornare alla vita normale

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, come sappiamo l'emergenza Covid-19 e le misure restrittive

Questo ha comportato, ovviamente, una drastica riduzione dei fatturati e una crisi di liquidità, che le società e le associazioni sportive hanno subito e i cui effetti negativi, purtroppo, si vedranno anche nei prossimi mesi, con prospettive molto preoccupanti per l'intero settore.

tuttavia innegabile come gran parte delle realtà attive in questo comparto, e specialmente quelle che operano a livello dilettantistico e locale, abbiano manifestato chiaramente il rischio di cessazione dell'attività, se non conosceranno in tempi brevi le modalità per rilanciare il settore. Parliamo di numeri davvero importanti, signor Ministro, che lei conosce bene. Questo significa soprattutto far venire meno un'attività fondamentale nei territori, quella cioè dello sport di base: pensiamo a quanto hanno sofferto i nostri figli in questi mesi, con la chiusura delle scuole con lo sport che non si poteva praticare. Questo è anche uno dei motivi per cui come Italia Viva abbiamo fatto una proposta, sia a lei che al ministro Azzolina: le palestre delle scuole devono rimanere ad uso esclusivo dello sport per i nostri figli, così come devono rimanere anche ad uso delle società e delle associazioni

di molte forze politiche, compresa Italia Viva, c'era la necessità di avere questi incentivi fiscali, proprio per far fronte all'emergenza, visto tanti sponsor territoriali sono in difficoltà, mentre le aziende in questo momento potrebbero ancora aiutare le società e le associazioni sportive nei territori. Questo credito di imposta è dunque per noi fondamentale, così come richiesto

che ha già avviato il tavolo, sia con la maggioranza che con la minoranza. Si toccheranno aspetti fondamentali per il mondo dello sport e noi vogliamo

Noi siamo in grado di soddisfare tutte le richieste, quindi, già dalla fine di questa settimana, partiranno i bonifici nei confronti di tutte le ASD e di tutte le SSD che hanno fatto richiesta. A volte sono richieste di 1.000 euro, a volte di 11.000 euro: ognuno ha documentato il tipo di difficoltà che ha avuto durante il periodo di pandemia e riceverà il sostegno proprio perché da parte mia, così come di tutto il Governo, c'è la convinzione che il tessuto sociale e culturale, che vede protagoniste molte

come recuperare anche tutte le risorse necessarie per la sanificazione continua degli ambienti e delle palestre scolastiche che di giorno potrebbero talvolta, in alcuni casi e in alcune Regioni, essere utilizzate per l'attività scolastica. Anche in questo caso il Ministero dello sport prevedrà un Fondo *ad hoc* per aiutare tutte le scuole ad avere le le risorse necessarie per garantire la sanificazione delle palestre, in modo che esse possano essere utilizzate, nella stessa giornata, sia per le attività scolastiche sia, poi, per le attività sportive. Per quel che riguarda il credito d'imposta, purtroppo anche nell'esame parlamentare del decreto-legge non è stato possibile inserire nulla

la delegazione di Italia Viva, che poi la stessa delegazione ha ritenuto di annullare, avendo bisogno di maggiore tempo per approfondire il testo. Siamo a disposizione e appena la delegazione di Italia Viva sarà pronta con l'approfondimento del testo, incontreremo. Sono d'accordo con lei: l'autonomia dello sport va salvaguardata e la politica deve rimanere fuori dallo sport. Questo è molto importante: la politica deve farsi interprete dei bisogni del mondo dello sport e non delle singole persone. Questo è molto importante, è un richiamo che accetto volentieri e

della legge delega, non c'è stato nessun problema da parte di Italia Viva, se non quello di aver ricevuto, solo in forma cartacea, una bozza di 124 pagine, tre giorni prima della riunione prevista e quindi, chiaramente, abbiamo chiesto più tempo, come altri partiti di maggioranza - mi risulta lo abbia fatto anche il Partito Democratico e non solo - proprio per poter affrontare meglio questo tema e chiedere che ci sia una riunione di maggioranza e non degli incontri separati tra le forze politiche. Questa era la richiesta, dopodiché mi auguro veramente si faccia una riforma nel modo migliore possibile e seriamente: qui non ci sono attacchi o difese di singole persone o di singoli posti. Proprio perché vogliamo farla bene, la dobbiamo fare insieme,

riguarda, rimarrò a sua disposizione, come gli altri colleghi e colleghe, per poter lavorare assieme e avviare un tavolo davvero permanente di lavoro,

fatta al Parlamento sul fenomeno della tossicodipendenza in Italia a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. In essa si legge addirittura che i decessi legati al consumo di stupefacenti sono stati 334 (quindi il 12,8 per cento in più rispetto ai 296 dell'anno precedente), addirittura con una quota rilevante anche tra le donne *over*

temi della liberalizzazione delle droghe leggere o dell'educazione sessuale nelle scuole, sarebbe forse meglio cominciare a fare un po' di educazione a non utilizzare e a contrastare le droghe. Infatti, nella maggior parte dei casi - lo dice proprio Anna Rita Calavalle, che va nelle scuole a insegnare - i ragazzi non sanno assolutamente che cosa stanno per assumere.

senatore, desidero in premessa chiarire che tra le mie deleghe non rientra specificamente il coordinamento delle politiche antidroga, materia che è rimasta in capo al Presidente del Consiglio dei ministri insieme a disabilità e protezione civile. Quindi, anche le azioni del dipartimento per le politiche antidroga del Governo, che pure esiste, non afferiscono in alcun modo al mio indirizzo politico, né sono dal mio Ministero vigilate. Fatta questa breve premessa e avendo però ritenuto il Senato che fossi io a dover riferire sull'interrogazione in discussione, fornisco alcuni elementi di informazione e valutazione rispetto a quanto è stato chiesto. Il dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ha in atto un piano di contrasto alle droghe che investe sui giovani attraverso azioni di prevenzione mirate. Dopo aver realizzato in passato campagne di informazione sulle droghe rivolte alla popolazione in generale, negli ultimi anni sono state promosse azioni di prevenzione sul territorio rivolte a *target* specifici e più vulnerabili, quali i giovani, che mirano a sviluppare azioni di sensibilizzazione e informazione di genitori, educatori e insegnanti. Sono in corso attività sul fenomeno dell'incidentalità stradale alcol-droga correlata alla prevenzione delle dipendenze, nonché attività sul territorio, anche d'intesa con tutte le Forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri e altre, per sensibilizzare sul fenomeno della compravendita da parte dei giovani delle sostanze stupefacenti, soprattutto *via* *web*; iniziative alle quali in parte abbiamo contribuito anche noi come Dipartimento per le politiche giovanili e Servizio civile universale. In modo particolare, con riferimento anche ad una proposta emendativa che era stata avanzata e non accolta in sede di conversione del decreto rilancio, alla quale anche adesso si faceva riferimento, l'obiettivo della stessa proposta era quello di implementare la filiera agroalimentare della canapa, settore che non è rimasto indenne dalla crisi economica conseguente all'emergenza Covid-19. Con la citata proposta emendativa, si introduceva inoltre la necessaria specificazione volta a stabilire che ciò che è consentito produrre dalle qualità di canapa certificata di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. del 2016, analogamente a quanto previsto per le piante, non rientrava nel contesto disciplinatorio del testo unico degli stupefacenti, di cui al decreto del tale riguardo, in generale, in merito al dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere, ritengo che la delicata questione dovrebbe essere rimessa al democratico confronto parlamentare tra tutte le forze politiche - come veniva ricordato anche all'inizio dall'interrogante - confronto rispetto al quale il Governo non mancherà certamente di intervenire in maniera costruttiva. che, per quello che riguarda il senso della partecipazione, il protagonismo, ma anche il livello educativo al quale lei faceva riferimento, con un piano che preveda il più possibile il coinvolgimento dei giovani, che è una parte che afferisce alle mie idee, le posso assicurare che da quando ho questa delega, che conservo anche dalla precedente esperienza governativa, la mia costante azione quotidiana

un'altra interrogazione così poi, in base ai numeri, vedremo se le politiche di prevenzione vengono poste in essere davvero. Non vedo tutto il grande coinvolgimento del mondo della scuola, al di là della della questione del Covid, che chiaramente ha tenuto lontani gli alunni dagli istituti scolastici. Non vedo la grandissima attenzione anche mediatica, culturale, di protagonismo per cercare di fare in modo che i ragazzi capiscano

Si stima che annualmente si spendono 4,4 miliardi di euro per le sostanze stupefacenti, derubricate a mere droghe leggere. Non a caso, il 58 per cento delle operazioni antidroga e il 96 per cento dei quantitativi sequestrati,

le giovani generazioni, perché di solito i giovani sono quelli che propongono i cambiamenti, le rivoluzioni che, nella storia, hanno sempre fatto i grandi passi. Consentendo loro di utilizzare droghe più

politiche o crede nei complotti. Proprio per questo motivo ritorneremo su questo tema e la reinterrogheremo. A questo punto rivolgeremo l'interrogazione al presidente Conte, con la speranza che venga ogni tanto anche a farsi interrogare - come diceva che avrebbe fatto, visto che voleva parlamentarizzare tutto in modo tale che avremo anche qualche risposta sul fronte delle politiche attive dal Ministero - come lei dice - direttamente competente.

ieri alle prime luci dell'alba, sulla superstrada che collega Barletta ad Andria, è avvenuto un terribile incidente. Un furgone ha travolto una bicicletta elettrica con tre ragazzi di Barletta a bordo:

La comunità cittadina è fortemente scossa dall'accaduto. Innanzitutto voglio esprimere il mio turbamento per la prematura scomparsa e la mia vicinanza ai familiari dei ragazzi. Condivido con tutto il mio cuore il dolore straziante che improvvisamente li ha trafitti. Come prassi, è intervenuta la magistratura e sono in corso le indagini del caso per accertare la dinamica dell'incidente, le circostanze e le eventuali responsabilità. Aspettando con fiducia il loro esito, penso che l'accaduto debba indurre seri interrogativi a noi legislatori, ai responsabili dell'ordine pubblico e a tutti i cittadini. Le biciclette elettriche hanno sicuramente una fondamentale importanza ecologica e vanno incentivate per favorire la mobilità sostenibile, soprattutto quella urbana; ma occorre costruirle con *standard* di sicurezza elevati e con un limitatore di velocità non modificabile. Le *e-bike*, oltre all'osservanza del nuovo codice della strada modificato dall'articolo 229 del decreto-legge rilancio, dovrebbero sottostare a norme di sicurezza stradale più rigide: casco e luci obbligatorie, patentino, targa. Altrettanto costanti e rigidi dovrebbero essere i controlli delle Forze dell'ordine. Sono indispensabili interventi strutturali per costruire corsie preferenziali per bici, piste ciclabili urbane secondo una rete efficiente (per evitare frequenti uscite ed entrate dalle corsie), corsie riservate extraurbane, ciclovie. L'educazione civica e stradale deve essere martellante e diffusa in tutte le agenzie educative, per indurre i ragazzi a comportamenti civici e consapevoli. Di certo nulla può restituirci le vite perdute, né lenire il dolore, ma abbiamo il dovere di agire, per evitare nel futuro tragedie disperate similari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo oggi la parola per porre all'attenzione di quest'Aula quanto successo ieri a Palermo. Si è abbattuto sulla città un violento nubifragio estivo. Il cambiamento climatico è una realtà e sta provocando impatti e fenomeni di frequenza e intensità mai visti nella storia umana; e con essi sofferenze, perdite di vite, sconvolgimento degli ecosistemi e della ricchezza di biodiversità che sostengono la nostra vita. Bombe d'acqua, incendi, disboscamento, dissesto idrogeologico, innalzamento della temperatura, inquinamento ambientale e marittimo in particolare stanno creando non pochi problemi a tutto il pianeta. Sul capoluogo siciliano è caduta una grande quantità di pioggia, che ha allagato in pochi minuti alcune zone della città. In due ore la bomba d'acqua che si è abbattuta su Palermo ha allagato i sottopassaggi in viale della Regione Siciliana, bloccando numerose auto che transitavano. Ricordo che il viale della Regione Siciliana è una grande arteria, molto frequentata, che collega le autostrade di Trapani e Catania. Si è trattato di un evento eccezionale, con pochi precedenti; di un forte nubifragio che ha scaricato un'enorme quantità d'acqua di pioggia), con precipitazioni intense e violente, in uno spazio temporale di due ore, mettendo in ginocchio la città di Palermo. Le condizioni meteo sono ormai fortemente condizionate dai processi di antropizzazione che hanno cambiato il clima e l'ambiente. Le strade interne si sono trasformate in fiumi; abbiamo assistito ad immagini incredibilmente drammatiche: macchine sommerse e persone costrette ad uscire dagli abitacoli e a nuotare per mettersi in salvo. I Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno lavorato fin dalle prime ore pomeridiane e per tutta la notte e sono ancora sul posto, con le squadre speciali dei sommozzatori e con le idrovore, per verificare le macchine rimaste nell'acqua e nel fango alla ricerca di dispersi. stati gli interventi, anche per sgomberare case ed evacuare palazzi a rischio di crollo. E allora il primo ringraziamento va a tutta la macchina dei soccorsi, ai Vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e locale che, con coraggio e tempestività, hanno svolto i propri doveri prestando i soccorsi necessari e salvando dal peggio gli sfortunati cittadini che si trovavano a passare in quelle strade allagate. Questa mattina su Palermo splende il sole e sono più visibili gli effetti del disastro causato dalla fortissima pioggia. Il mio abbraccio va a tutti i palermitani, in attesa dei rilievi e delle indagini che appureranno eventuali responsabilità.